la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta Illustre Presidente, ho l'onore di comunicarLe, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletto Presidente. Firmato: Augusto Antonio Barbera». A nome mio e di tutta l'Assemblea, rivolgo al presidente Barbera, che ho sentito al telefono, anche i più cordiali auguri di buon lavoro.

consegnato il testo delle sue comunicazioni, che ha già reso alla Camera dei deputati, e questo la esime dall'illustrarle nuovamente. Avverto

ringrazio con il più vivo apprezzamento il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per una relazione che ci dà la prova di un'azione di Governo estremamente incisiva nel tracciare con pieno successo un cammino sicuro per l'Italia, un cammino sicuro in Europa e nel mondo. Ci troviamo di fronte un Consiglio europeo difficile, non privo di insidie. Il Presidente del Consiglio ha ritenuto di fornirci in sintesi le sue valutazioni sullo stato della trattativa sul Patto di stabilità ancora aperta, precisando quanto la posizione italiana sia chiara e rispettata a Bruxelles. Riconosciuti apprezzamenti sono giunti dall'Europa per i risultati ottenuti nella politica di bilancio, che garantisce stabilità, credibilità e coerenza del nostro Paese. La scadenza decisiva, come sappiamo, è il 31 dicembre: potrebbe andare oltre il negoziato rispetto al Consiglio europeo, come ha detto il Presidente del Consiglio, l'ipotesi di proseguire i lavori, ma è importante continuare a cercare di bilanciare le esigenze di disciplina fiscale con la flessibilità necessaria per affrontare le sfide economiche, rispettare la disciplina fiscale, ottenere credibilità e fiducia, garantire anticiclicità e i giusti incentivi per investimenti e riforme incentrate sulla crescita, che rispondano alle priorità europee condivise. Il punto di partenza riguarda i piani nazionali a medio termine, che dovranno costituire la base del dialogo con la Commissione: vengono fissati i parametri di salvaguardia, che potrebbero essere problematici, se non fossero considerati anche il contesto macroeconomico ed economico-sociale nel loro insieme e se non fossero considerati gli impegni assunti nell'ambito del PNRR. Ci sono quindi elementi positivi, frutto soprattutto del duro lavoro negoziale svolto in queste settimane dal Presidente del Consiglio, efficacemente coordinato dai ministri Giorgetti e Fitto.

non consideravano gli aspetti di *spillover* in negativo che tali misure di austerità avrebbero provocato. Ne siamo usciti soprattutto grazie alla flessibilità dimostrata dalla Banca centrale europea. I fronti ora aperti per l'Unione europea sono molteplici: è essenziale una *leadership* autorevole e riconosciuta come quella del presidente Meloni, che tenga fede ai valori comuni europei, alle alleanze internazionali e alle sfide che si prospettano. Oltre ai negoziati sul Patto di stabilità e crescita, vi sono quelli su migrazione e asilo, che hanno visto sempre l'Italia nell'ultimo anno attiva e propositiva e, nonostante le tante critiche espresse dall'opposizione per quanto riguarda gli aspetti economici, sulla terza e quarta rata del PNRR, l'Italia è riuscita a dare sostanza concreta con risultati straordinari. Il ministro Fitto ha spiegato che vi sono complessivamente 350 miliardi di risorse disponibili, se si considerano anche i fondi strutturali e di coesione. Lo stesso discorso vale sul ruolo riconosciuto all'Italia per l'immigrazione quanto alla politica estera, per la quale le nostre posizioni su Ucraina e Israele dimostrano quanto abbiamo tenuto fermi i principi e le regole dell'ordinamento internazionale.

che i trafficanti di esseri umani dovranno risarcire le loro vittime dei guadagni ottenuti grazie al loro sfruttamento. Questo indica quanto importante sia per la giurisprudenza europea il principio fondamentale di questa maggioranza in Parlamento di colpire la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani. *(Applausi)*. Questo è un elemento centrale che finalmente è stato acquisito, così come quello del controllo delle frontiere esterne dell'Unione è stato recepito ormai

in Italia, di chi entra legittimamente in Europa e di chi no e che comporta anche misure di rimpatrio molto più efficaci di quelle che sono state applicate sinora nel contesto europeo. Gli accordi con Tunisia e Albania sono visti anche in Europa come risultati positivi e ottimi punti di partenza e qui c'è sempre ancora la scelta del Governo di dialogare in un rapporto paritetico con i Paesi di transito quando questo dà i propri frutti, come il Presidente del Consiglio ha sottolineato nella sua relazione. L'Europa ci apprezza e domani al Consiglio europeo l'Italia si presenterà convinta delle sue ragioni, aperta, non certo vittima di propagande ideologizzate, ferma e decisa e non certo distratta da qualche gioco di carte. Le azioni che violano gravemente il diritto internazionale sono soprattutto oggi l'uso della forza che abbiamo visto moltiplicarsi negli ultimi due anni nel solco dell'aggressione criminale di Putin all'Ucraina. Dall'Ucraina al Medio Oriente fino all'Africa e al Mar della Cina, è l'uso della forza in violazione del diritto internazionale che sta imperando. Difendere l'Ucraina, esattamente come difendere Israele, significa difendere l'Europa. Troppi fingono ancora di non saperlo, ma senza i necessari aiuti americani ed europei, una sconfitta dell'Ucraina sarebbe solo l'inizio di una catastrofe. Il conflitto in Israele e il conflitto in Ucraina, contro l'Ucraina e contro Israele, sono mossi da un unico disegno revisionista e criminale. È per tale motivo che 134 parlamentari di 14 Parlamenti nazionali dell'Unione, tra i quali diversi italiani, hanno lanciato un accorato appello al Congresso americano affinché sia sbloccato il finanziamento richiesto dal presidente Biden in sostegno di Kiev. La capacità di difesa e di controffensiva ucraina è rallentata. Nell'ormai iniziata stagione invernale, gli attacchi russi sono deliberatamente mirati a distruggere risorse vitali per l'energia, l'alimentazione, gli ospedali e le scuole; attacchi effettuati con armi iraniane, nordcoreane e probabilmente anche transitate e fornite dalla Cina, armi che cercano di distruggere una Nazione e la sua identità. Ci sono purtroppo anche in Italia voci che tornano a inneggiare a Putin e alla sua possibile vittoria, quando nella realtà Putin è già stato sconfitto, diventando il vero *paria* della comunità internazionale. Le bombe russe hanno svegliato l'Occidente dal sonno della ragione che si era autoimposto. Abbiamo scoperto che la libertà non è né un frutto della natura, né un dono che cade dal cielo, ma anzi una continua conquista, una battaglia costante a cui l'Occidente non può presentarsi disarmato nello spirito e nella forza. La libertà è la condizione primaria, il concetto base di tutti i nostri valori occidentali, i valori universali. L'Europa comprende e apprezza la linea del Governo Meloni, che sin dal primo giorno sostiene con forza l'Ucraina, una linea ampiamente condivisa anche nei Parlamenti nazionali. Siamo di fronte a una guerra ibrida di disinformazione, di reti di influenza, di corruzione dei sistemi politici e delle istituzioni negli stessi Paesi fondatori dell'Unione europea e anche questo punto è presente nella risoluzione di maggioranza. Una questione che il Governo ha affermato ripetutamente nei vertici atlantici ed europei e ribadita nei giorni scorsi alla Conferenza interparlamentare dei Presidenti della Commissione per l'Unione europea di Madrid. Anche lì sono emerse aspettative, ma anche inquietudini sia per le decisioni del Consiglio europeo che per quelle del Congresso americano. Il controllo ucraino dello spazio aereo sull'intero territorio e la capacità di guerra elettronica sono sempre più due elementi fondamentali. Per Kiev è determinante poter acquisire una capacità di deterrenza anche tecnologica rispetto all'aggressore e di non essere più vittima di una rincorsa fra capacità tecnologiche russe e quelle che riesce - spesso troppo tardi - spesso ad avere. Zelensky ha dichiarato: la Russia spera in una sola cosa, che l'anno prossimo la solidarietà nel mondo libero collassi. È una questione di finanziamenti e aiuti, ma l'integrazione di Kiev nell'Unione europea è la chiave di volta per gli assetti europei e deve procedere speditamente. Fondamentale è anche la prospettiva di allargamento dell'Unione europea alla Moldavia e alla Georgia, ai Balcani occidentali e all'Albania: tutti Paesi che, come la presidente del Consiglio Meloni ha sempre ribadito, sono parte integrante dell'Europa. Altro punto cruciale per l'Europa è il sostegno senza se e senza ma a Israele e ai suoi valori. In questo caso entriamo nel discorso dell'antisemitismo, della brutalità genocidaria di Hamas il 7 ottobre scorso

siamo certi che lei e il Governo in Europa farete del vostro meglio

la restituzione del PNRR: miliardi e miliardi che vanno restituiti. Noi siamo l'unico Paese che ha un prestito così ingente da restituire.

Ti vengono condonati 20 miliardi di tasse, potremmo parlare di un condono di 20 miliardi l'anno. Questo è l'impatto di questi *bonus* fiscali sull'edilizia. È chiaro che con questi due macigni è tutto più complicato e il piano di rientro del debito è particolarmente difficile, però noi siamo fiduciosi perché sappiamo che il Governo ha questa consapevolezza. Faccio un altro esempio: pochi sanno che fu proprio il ministro Giorgetti a introdurre quella flessibilità nel pareggio di bilancio che consente di fare un minimo di manovra. Ebbene, se non ci fosse stato quell'intervento del ministro Giorgetti nella revisione delle regole costituzionali sul pareggio di bilancio, noi non avremmo flessibilità, saremmo a zero nel fare le leggi di bilancio. Ricordo che all'epoca il buon Giorgetti si beccò gli strali di una certa sinistra, articoli e critiche di Giavazzi e Alesina sul "Corrierone" per aver introdotto quella flessibilità. Meno male che c'è questa

semplice e giusto. Concludo con una nota positiva proprio su questo tema dei redditi. Recentemente, la presidente del Consiglio Meloni è stata sul Lago Maggiore, in una bellissima struttura. Non so se ha avuto modo di parlare con il titolare, ma i dipendenti di questa struttura hanno avuto un aumento di stipendio di 400 euro, tutti, dalla signora delle pulizie al cuoco, dal portiere al cameriere. Come mai sono stati dati 400 euro netti in più in busta paga a tutti?

Ebbene, aiutateci a diffondere questa buona prassi, perché la possibilità concreta di aumentare gli stipendi, anche in modalità come quelle che ho

sappiamo che quello di giovedì e venerdì sarà un Consiglio europeo molto importante non solo per i temi all'ordine del giorno, ma anche per il momento storico estremamente particolare.

che è molto cara a tutti noi e a me in particolare, del presidente Draghi in treno con Macron e Scholz. Quel treno era diretto in Ucraina.

non ancora propriamente in Europa - attaccato e massacrato dalla politica di invasione e di aggressione di Putin.

Lei quella foto non la può vantare o portare a sé, perché le foto che lei ha non sono così simboliche come quella di quel momento. *(Commenti).* Ripeto, è l'Europa che cerca di prendere per mano l'Ucraina, che oggi ci chiede di essere Europa e che in questo Consiglio europeo avrà un ruolo da protagonista in questa direzione. Lei purtroppo ha tante foto con Orban, che è colui che non voleva neppure che il tema dell'Ucraina entrasse nell'ordine del giorno del Consiglio europeo che ha scritto una lettera non più tardi di una settimana fa chiedendo che venisse tolta l'analisi sull'Ucraina dal Consiglio europeo. Capisco, colleghi, che questa cosa sia molto imbarazzante per voi, ma ognuno si sceglie i compagni di viaggio che vuole. Diciamo che comprendiamo benissimo il vostro imbarazzo, ma io cerco di capire anche l'imbarazzo dei colleghi che con me sono nella

quello spiraglio, quelle alleanze e quei ponti per riuscire a essere inseriti davvero in Europa e far partire quel processo. Sappiamo che il Consiglio

per esponenti politici, per capi, come Orban, che questa linea non la vogliono e la sconfessano. Un minimo di vergogna o di imbarazzo secondo me c'è. Non voglio trascurare però anche un'altra questione, che è quella che stanno vivendo i Paesi dei Balcani. Sappiamo che in questo Consiglio europeo ci sono nuove raccomandazioni, in modo particolare per la Serbia e per la per la Bosnia-Erzegovina. Tali raccomandazioni mettono tutte al centro le scelte in politica estera, chiedendo a questi Paesi una sorta di coerenza nella politica estera, legata poi anche agli amici che si frequentano. la richiesta? Un allineamento con la politica estera dell'Unione europea, comprese le misure restrittive e le dichiarazioni sulla Russia. È come se l'Europa chiedesse a tutti - e lo ribadisse - che per entrare a far parte dell'Unione europea si devono condividere gli stessi valori, la stessa visione di mondo e la stessa concezione di Stato di diritto. È difficile pensare che chi non ha questa concezione possa essere un buon alleato per l'Italia anche in queste battaglie giuste e sacrosante *(Applausi)*, perché fanno perdere la reputazione. Fanno perdere la reputazione! È per questo che io ritorno sul tema delle compagnie, dei compagni di viaggio, delle amicizie e delle frequentazioni. Presidente Meloni, io so che

alla discrasia tra le cose che per esempio la sua forza politica e lei avete detto durante le campagne elettorali o negli anni passati e quelle che state facendo. Non ho intenzione di di ripeterle perché siete più svelti voi di me, basta googlare per vedere le dichiarazioni che avete fatto negli anni nei confronti dell'Europa. Tutto rimane lì, perché purtroppo i *social* non salvano più nessuno. Presidente, lei è bravissima - non

nelle repliche perché, se andiamo a vedere invece i tempi del suo Governo (sono uscita ora dalla Commissione bilancio), vorrei stendere un velo pietoso.

infatti come farà a sedersi a fianco a Sanchez dopo le parole che il suo amico Abascal ha pronunciato contro di lui. Nonostante queste parole, lei continua a pensare che sia corretto invitarlo ad Atreju. Vorrei ricordare qui quali sono le parole che sono state dette e l'invito a essere messo a testa in giù. vi foste nascosti dietro un ago. Non entriamo - ho concluso, Presidente - nelle vicende di un altro Paese. Peccato che il *leader* di questo Paese, della Spagna, stia lavorando a fianco del nostro per un Patto di stabilità più giusto. Evidentemente vi trovate meglio, invece, a sedervi a fianco a Wilders, che sostiene che all'Italia non andrebbe dato neanche un centesimo. Ma lo ripeto: le questioni, Presidente, di coerenza riguardano i compagni di viaggio che uno decide di scegliersi. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, il prossimo Consiglio europeo sarà uno dei più impegnativi. L'avvicinarsi della scadenza elettorale del giugno prossimo sta determinando l'intensificarsi dei negoziati sui tanti dossier legislativi all'attenzione del legislatore europeo, come quello chiuso da poco sull'intelligenza artificiale, sulle case *green* e sulle materie prime critiche. Molti altri sono in corso di finalizzazione e, tra questi, sono importanti per il nostro Paese quello sul quadro finanziario pluriennale, quello sul Patto per la migrazione e l'asilo e quello sul Patto di stabilità e crescita. Dunque i temi all'ordine del giorno sono tanti. L'aggravarsi della situazione a Gaza è sotto gli occhi di tutti e dobbiamo lavorare affinché si arrivi quanto prima ad una soluzione a lungo termine per la stabilizzazione dell'area, senza tuttavia dimenticare i vili attacchi terroristici contro Israele commessi da Hamas e ribadendo il diritto dello Stato di Israele alla propria esistenza, sicurezza e difesa, la cui legittimità sul piano del diritto internazionale, per quanto da qualcuno contestata, è evidente. La situazione è difficile e i morti sarebbero quasi 20.000. Con la risoluzione che voteremo ribadiamo l'impegno dell'Italia nel fronteggiare l'emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, già dimostrato mediante l'invio in questo contesto di materiale umanitario dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi e dalla nave ospedale "Vulcano", per la cura in particolare dei minori feriti a Gaza. È necessaria una presa di posizione forte del Consiglio europeo e auspichiamo una soluzione sulla scia di quanto già messo in campo dal nostro Governo. C'è poi la questione dell'allargamento dell'Unione, con la possibile apertura dei negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldova e con la concessione dello *status* di Paese candidato alla Georgia. Senatrice Malpezzi, il Governo italiano sta facendo la sua parte, glielo assicuriamo. sono un senatore del Mezzogiorno, dove le politiche di coesione europee pesano molto nel bilancio complessivo e dove la politica agricola comune pesa molto sul reddito di tante famiglie. Dovremmo quindi essere preoccupati per l'ingresso di Stati che inevitabilmente, per la loro dimensione e popolazione, comporteranno una possibile penalizzazione per le politiche tradizionali europee. Ma c'è una dimensione politica che non possiamo dimenticare; c'è un nostro impegno, assunto più volte in quest'Aula, per dare un segnale di incoraggiamento al popolo ucraino, che sta subendo una brutale aggressione da quasi due anni. Per questo siamo assolutamente a favore del loro ingresso nell'Unione e dell'apertura dei negoziati di adesione, essendo consapevoli delle riforme che necessariamente l'Unione europea dovrà mettere in campo per accogliere i nuovi membri. Fare il possibile per garantire questo risultato è un punto di coerenza che è la cifra politica del Governo. C'è poi la questione della riforma del Patto di stabilità, dovrebbe essere un trampolino per la prosperità di ogni Nazione e non solo un insieme di regole rigide. Come più volte ha ribadito il ministro Fitto, il Patto, oltre a garantire la stabilità, serve anche per consentire la crescita. Per questo l'intesa risulta essenziale, proprio per evitare il ritorno delle regole di bilancio che hanno disciplinato i conti pubblici europei fino allo scoppio della pandemia di Covid. A tal proposito, Presidente, siamo soddisfatti che - come lei ha annunciato - la bozza di accordo delle ultime ore sul Patto di stabilità vada a riconoscere di fatto la posizione portata avanti dall'Italia in sede europea, secondo cui vi debbono essere regole di bilancio che consentano di attuare le politiche dell'Unione. In questo senso, gli obiettivi di riduzione del rapporto *deficit*-PIL dovranno tenere conto degli investimenti per la difesa e la transizione verde e digitale. Abbiamo da sempre contrastato le vecchie regole, proprio perché mancava questa logica consequenzialità di coerenza, che ci chiedevano un'austerità complessiva, quando invece era necessario diversificare gli approcci tra gli Stati membri. Non ha senso, dunque, imporre nuovamente dei vincoli che, già in occasione della pandemia, hanno dimostrato tutti i loro limiti e infatti erano stati sospesi. La storia è andata avanti: non possiamo tornare indietro. L'obiettivo del Patto di stabilità non può e non deve essere limitare, ma deve garantire la resilienza delle economie nazionali, permettendo loro di crescere in modo sostenibile. Quindi, presidente Meloni, massima vigilanza e pieno sostegno alla sua azione, tesa a evitare rigidità e meccanismi automatici che, pur mirando alla riduzione del debito, non tengano conto dei necessari meccanismi di crescita, danneggiando, di conseguenza, la nostra economia. Confidiamo in un accordo dignitoso nell'imminente riunione Ecofin entro la fine dell'anno. ultimo punto, signor Presidente del Consiglio: si sta lavorando in sede europea a possibili riforme e a possibili modifiche dei trattati. Credo sia importante, anche per l'Italia, offrire il proprio contributo al dibattito sulle riforme, per individuare le soluzioni più adeguate in materia di politiche, risorse e, in prospettiva, meccanismi e assetti istituzionali, affinché l'Unione sia pienamente all'altezza delle sue ambizioni e del suo ruolo nel contesto globale. Come ha anche ribadito il nostro Presidente della Repubblica, il 2024 sarà caratterizzato da un grande esercizio di democrazia: il popolo europeo sarà chiamato a eleggere il Parlamento d'Europa, massimo organismo rappresentativo delle volontà dei cittadini e del Continente. Ecco, iniziamo dal prossimo Consiglio europeo, per poi arrivare a portare a compimento le tante riforme che i nostri cittadini attendono da tempo. Presidente Meloni, l'Italia e l'Europa si fidano di lei, confidano in lei. Tutti in quest'Aula dovrebbero sperare nel raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si prefigge. La politica non si può dividere sugli interessi della Nazione e neppure su una fotografia, senatrice Malpezzi. Signor Presidente, chiudo con una riflessione. Grandi uomini come De Gaulle ci hanno insegnato che l'Europa deve essere non un super-Stato, bensì una comunità di Nazioni sovrane, rispettose delle proprie tradizioni e culture, ma che vanno avanti, unite nelle proprie diversità, sul lungo cammino della storia. Ecco, adesso tocca a noi percorrere un pezzo di quel cammino, consci della responsabilità che abbiamo, ma pronti a raccogliere anche questa sfida. *(Applausi)*.

Se volessimo utilizzare un'immagine retorica un po' datata, potremmo dire che «uno spettro si aggira per l'Europa». Non è quello del 1848, ovviamente, ma è quello del disimpegno e del benaltrismo e, in alcuni casi, anche quello del cinismo. Uno spettro che si insinua in questo che è stato definito il tempo dei sonnambuli. È la definizione della società italiana secondo il Censis; è il vocabolo per descrivere la classe dirigente della Belle époque, che ci condusse alla Prima guerra mondiale, secondo un bel libro di Christopher Clark; ma è anche la definizione con la quale Liz Cheney, la figlia del vice presidente di George Walker Bush, ha definito gli americani che si apprestano ad appoggiare Trump. Insomma, la domanda, signora presidente Meloni, è semplice e precisa: il Governo, nell'era del sonnambulismo, da che parte state? E, soprattutto, dove volete portare l'Italia? In Europa, infatti, ci sono *leadership* spregiudicate, che stanno sfruttando la vicenda dell'Ucraina per insinuare l'antica logica dell'*appeasement* di chamberlainiana memoria. La domanda che vorremmo fare è la seguente: quale idea d'Italia, quale idea d'Europa vorrete rappresentare a questo Consiglio europeo? L'idea di Wilders, nemico storico dell'Italia quanto sodale stretto del suo vice premier Salvini, oppure l'idea del suo amico Abascal, che lei si appresta ad ospitare, che vuole appendere il *Premier* spagnolo a testa in giù? Oppure, ancora, quella del suo amico Orban, che non vuole Kiev in Europa e si mette alla testa della fronda sovranista, che fa sorridere il Cremlino? Lei ieri si è innervosita alla Camera dicendo che non si fa la politica estera con una foto. Sarà, ma in ogni caso i suoi *selfie* in riva al Danubio con Orban nelle cancellerie europee non li dimenticano. E la verità di quella foto che lei non digerisce, quella del treno per Kiev, non stava tanto nell'immagine, quanto nel valore simbolico da essa trasmessa: il valore del prestigio dell'Italia che viaggiava, *primus inter pares*, tra i grandi per dare solidarietà a un popolo aggredito. *(Applausi)*. Quel prestigio - mi creda, signora Presidente - per lei e per il Governo, è ancora ben lungi dall'essere conseguito e per raggiungerlo non si dimentichi che diritto e giustizia, in latino, nascono dalla medesima desinenza: quindi, agisca di conseguenza senza ambiguità e, se possibile, anche senza troppe nevrosi.

ho apprezzato le sue comunicazioni, così come apprezzo in generale la politica estera condotta da lei e dal vice presidente Tajani e apprezzo molto l'opera sul fronte europeo dei ministri Giorgetti e Fitto: un'opera tenace ed efficace. Sul tavolo del Consiglio europeo e anche dell'Ecofin c'è un mosaico con molte tessere e lei, nelle sue comunicazioni, le ha menzionate tutte. Su alcune di esse esprimerò la mia opinione telegraficamente e di questo mi scuso. Allargamento è un imperativo storico, certo, ma mai e poi mai in passato si è parlato di allargamento nell'Unione europea in modo così superficiale, impreparato, sbrigativo e pericoloso. pericoloso sia perché non si sono fatti passi avanti decenti, né c'è una prospettiva chiara per farli, per quanto riguarda la modifica delle regole di funzionamento interne all'Unione, e anche perché non abbiamo minimamente preparato in nessun Paese le opinioni pubbliche a un allargamento di tanta portata. Il lavoro risulterà perfettamente inutile, con tante illusioni create e poi cassate, se le opinioni pubbliche in quei Paesi dove il *referendum* è necessario per i trattati di adesione diranno di no. Quindi, pensateci bene. Per dare maggiore snellezza di funzionamento all'allargamento dell'Europa, un giorno che sarà allargata, naturalmente è importante modificare le regole. Nell'ultima occasione ci siamo intrattenuti sul tema del passaggio alla maggioranza qualificata nelle decisioni di politica estera. Come lei sa, il suo ministro e vice presidente Tajani ha sottoscritto un'iniziativa di origine tedesca che riguarda tanti altri Paesi per passare alla maggioranza qualificata in politica estera. Lei è stata un po' *dismissing* su questo punto l'altra volta; la pregherei di riconsiderarlo, perché l'Italia ha molto bisogno di una politica estera per la quale lei, tra l'altro, dimostra molto gusto e attitudine, e avere il moltiplicatore europeo al suo fianco sarebbe importante. Spero che non si lascerà guidare nell'avere una posizione critica verso la maggioranza qualificata, anziché l'unanimità in politica estera, da alcuni membri della sua coalizione di Governo e da alcuni partiti facenti parte del Gruppo politico che lei presiede in Europa. qui deve rispondere dell'interesse nazionale italiano. E, comunque, sull'allargamento mi permetto di richiamare l'articolo di Maurizio Ferrera nel «Corriere della Sera» di oggi che dà una prospettiva concreta. Sul Patto di stabilità, esso non è accettabile. Lei l'ha un po' fatto capire, ma vorrei sottolinearlo: questo Patto di stabilità non è accettabile, non tanto per l'Italia, ma per l'Europa. È un'Europa con lo specchietto retrovisore quella che viene fuori da questo Patto di stabilità. Era questa l'occasione per dare molto più spazio a seri investimenti pubblici. Qualcuno si è divertito a dire: «Ah, Monti adesso cambia opinione a favore degli investimenti pubblici?». La memoria è corta, ma fin dal 1997, quando il Patto di stabilità è stato confezionato dalla Commissione europea, di cui ero membro, ma non competente per questa materia, ho insistito per uno spazio agli investimenti pubblici,

In Italia alcuni Governi ci hanno presentato come un successo nazionale l'aver ottenuto tanti miliardi di flessibilità, magari riferita filosoficamente agli investimenti, ma spesa in *bonus* a scopo elettorale. Non è questo che noi e lei vogliamo dal Patto di stabilità. Quindi sarei non minimamente scandalizzato, ma abbastanza lieto, se lei, in caso di necessità, usasse il veto sul Patto di stabilità, ma non può andare là piena di veti. Sul MES inviterei pertanto a una riconsiderazione: cerchiamo di essere seri. Anzitutto - e questo prescinde del tutto dalla riforma del MES - si ricorda che si era parlato del MES sanitario? Ebbene,

e quella è una possibilità molto ricca di prendere finanziamenti a scopo sanitario. Lei, che è maestra nella politica, mi insegna che mai in un sistema parlamentare la spesa sanitaria sarà finanziata adeguatamente, perché non è quella che ha dietro i gruppi di pressione più forti.

ossia portare nelle due Aule di Montecitorio e Palazzo Madama un disegno di legge di ratifica con l'ulteriore condizione che, se mai il Governo o i Governi dovessero utilizzare gli strumenti previsti dal MES,

luogo, a differenza di molti Governi precedenti, non svende l'Italia. Gliene siamo grati, ma queste sono due cose fondamentali, di primaria grandezza, di cui rallegrarsi. Immagino, Presidente, che ai suoi occhi l'ultimo Governo che ha reso orgogliosi gli italiani e non ha svenduto l'Italia sia quello di cui ha fatto parte nel periodo 2008-2011, l'ultimo composto dalle stesse forze politiche che compongono oggi la sua maggioranza. Quel Governo si dimise nel novembre 2011, dopo aver accettato di eseguire tutte le raccomandazioni elencate in una lettera altamente irrituale del Presidente della Banca centrale e del Governatore della Banca d'Italia. La maggioranza si ruppe in particolare perché una delle componenti, la Lega, non voleva accettare ciò che le altre avrebbero accettato, e cioè la riforma delle pensioni. Tra parentesi, sono molto lieto di quello che ho ascoltato ieri: dev'esserci stato nel frattempo un intervento provvidenziale perché, dopo quei momenti scandalosi di riforma delle pensioni in passato, lei ha scritto - e credo che sia vero - che oggi l'Italia ha uno dei sistemi pensionistici più sostenibili. Magari tutti gli italiani sono orgogliosi, anzi certamente sono orgogliosi del suo Governo e di lei, glielo auguro. Tenga presente che non necessariamente tutti gli italiani sono sempre completamente smemorati.

Signor Presidente, vorrei prima di tutto ringraziare la Presidente del Consiglio perché quando ci si presenta davanti al Parlamento in vista di un delicatissimo Consiglio europeo, importante non solo per le sorti dell'Unione europea, ma soprattutto dell'Italia, sarebbe fin troppo facile cadere nel tranello della politica degli annunci. Ne abbiamo visti di *leader* far finta di mostrare i muscoli in quest'Aula per poi nascondersi a Bruxelles, dove in passato ci si presentava con la sindrome di Stoccolma nella speranza di ottenere qualche concessione. Da quando si è insediato, malgrado la diffidenza, questo Governo invece ha avuto la capacità di far sentire le ragioni dell'Italia. l'ha fatto non con arroganza ma con serietà, dimostrando capacità di mediazione, con proposte concrete e ragionevoli, che rappresentano la realtà italiana in una dimensione europea. Ed è un fatto che alla riunione Ecofin per la modifica del Patto di stabilità si terrà nel dovuto conto la posizione dell'Italia per arrivare a un accordo prima della fine dell'anno. Non ci accontentiamo di un compromesso al ribasso. Quello del ministro Giorgetti e del Governo è un lavoro importante, che finalmente ha aperto per la prima volta la strada alla possibilità che venga riconosciuto lo sforzo di chi fa investimenti, soprattutto se questi investimenti sono collegati alle politiche dell'Unione europea, a partire dalla transizione *green* fino alla transizione digitale e spese per la difesa, che ovviamente in questo quadro geopolitico sono particolarmente importanti. Il nuovo patto non può essere il ripristino delle vecchie regole, non si può tornare all'austerità e servono norme espansive che riconoscano gli investimenti. Lo voglio dire forte e chiaro: non può essere l'Europa tutta a pagare le contraddizioni delle scelte politiche tedesche. *(Applausi)*. Forza Italia - come ha sempre sostenuto - non è pregiudizialmente contraria alla ratifica, ha delle riserve - questo sì - perché sono cambiati i tempi e le condizioni, perché va modificato il suo regolamento in un quadro di insieme macroeconomico e perché è profondamente sbagliato che la sua *governance* non sia sottoposta ad alcun controllo. In questo dibattito, a tratti surreale, ho sentito dire davvero di tutto. E allora, amici della sinistra, mettetevi d'accordo: o il MES serve a salvare i bilanci in caso di crisi finanziaria o difficoltà di collocamento dei titoli nazionali sul mercato - nessuno di questi due casi riguarda il nostro Paese, per fortuna - oppure serve per finanziare la spesa corrente. Questa confusione dimostra che la vostra è solo propaganda. E, invece, è importante che la ratifica del MES rimanga agganciata al negoziato più ampio sulla *governance* economica. E ancora più importante sarebbe sostenere il Governo nel chiedere che la BCE, che finora ha portato avanti una politica miope, dannosa per cittadini e imprese, abbassi i tassi - come ha dichiarato il ministro Tajani - e li abbassi ora che l'inflazione è scesa: risparmieremmo soldi da destinare alla sanità, alle pensioni, al salario minimo, alle tante mirabolanti idee che vi vengono in mente soltanto ora, dopo aver governato dieci anni. Che peccato! Intanto, le risorse per sostenere la crescita le stiamo ricavando dalla rimodulazione del PNRR. Soltanto che pensare di cambiarlo era impossibile, era da irresponsabili. Ebbene, i vostri scenari apocalittici si sono rivelati totalmente infondati. E, grazie all'incessante lavoro del ministro Fitto e degli altri Ministeri coinvolti, oggi il nostro è il primo Paese europeo a ricevere la quarta rata e il primo a essere pronto a presentare gli obiettivi della quinta. Non solo: grazie alla rimodulazione si liberano risorse importanti per le infrastrutture, per il sostegno della competitività delle nostre imprese. Noi siamo sempre rimasti aperti al confronto, ai suggerimenti, ai contributi. Voi, invece, avete preferito usare cinicamente come scudi umani i bambini e i malati, sostenendo falsamente che asili nido e ospedali, compresi quelli di prossimità, sarebbero stati penalizzati dalla modifica del PNRR. Ebbene, siete stati ancora una volta smentiti dai fatti. *(Applausi)*. Questa si chiama serietà e questi si chiamano risultati. risultati. Un altro importante risultato è stata la sacrosanta decisione di non rinnovare il *memorandum* sulla Via della seta, anche perché siamo l'unico Paese del G7 e dell'Europa occidentale ad averlo sottoscritto. Anche in questo caso il Governo è stato capace di garantire un atterraggio morbido, non provocando una rottura brusca o l'interruzione dei rapporti commerciali con la Cina, anzi dialogando per proseguire nei rapporti commerciali con un nuovo e più proficuo rapporto, senza essere egemonizzati dall'economia asiatica. Ancora una volta il Governo ha dimostrato di avere la schiena dritta e idee chiare; di avere una posizione politica ben precisa che riesce ampiamente ad avere pari dignità nei consessi europei e mondiali, nonché la credibilità che ci permette di far valere a Bruxelles la nostra posizione sull'importanza di guardare ai Balcani occidentali, non solo come regione regione di transito dei flussi migratori, con quel rischio di infiltrazioni nel nostro Paese di possibili terroristi islamici che ha portato alla temporanea sospensione degli accordi di Schengen, ma come opportunità. È giusto e auspicabile anche l'allargamento a Est dell'Unione europea per l'Ucraina, che ha diritto al suo futuro europeo. Dobbiamo però tenere in considerazione che l'ingresso potenziale tra alcuni anni di un Paese così grande in una condizione post bellica potrebbe comportare un impatto molto consistente rispetto a due partite storicamente molto importanti per l'Italia: la politica agricola comune (PAC) e la politica di coesione. Questo ci porta a dover studiare investimenti e strumenti giusti per far fronte a questa sfida, senza far venir meno il nostro sostegno a Kiev.

Tifate contro l'Italia, ma state raccogliendo soltanto delusioni: il PIL del 2023 è cresciuto più della media europea; lo *spread* è in calo; la Borsa vola;

primo Stato dell'Unione europea ad avere via libera sulla quarta rata del PNRR. Neanche il prezzo della benzina vi dà soddisfazioni, visto che è sceso a 1,70 euro. Con il centrodestra al Governo, come vedete, l'Italia è tornata forte e credibile, perché il Governo non naviga a vista, ma ha idee, prospettive, proposte e credibilità per realizzarle. Non è rischiare, non è affrontare il mare al buio e senza bussola: significa saper dove andare, aver chiaro in mente il nostro orizzonte politico e lei, Presidente del Consiglio, con l'intero Governo, lo sta dimostrando davvero a tutta l'Italia.

Presidente del Consiglio Meloni, ci rivediamo puntualmente ogni volta che c'è in programma un Consiglio europeo. Ora i temi in agenda sono veramente tanti, ma proverò a puntare l'attenzione su alcuni punti. A me dispiace non vedere presenti alcuni Ministri, in particolare il ministro Giorgetti, visto che il tema legato al Patto di stabilità sarà uno di quelli nodali nell'agenda

La vedo molto attenta, sta prendendo appunti, magari già si sta portando avanti con i lavori, come è giusto che sia. Io la ringrazio per l'attenzione, ma sarebbe opportuna la presenza dei ministri interessati.

si rivolga a me, per favore. per cercare di difendere l'indifendibile, in quanto voi con la manovra di bilancio avete dimostrato qual è il vostro approccio, in che modo pensate di rilanciare la Nazione, e cioè con l'austerità. *(Applausi)*. L'Istat vi ha bocciato sonoramente.

politica austera che sta portando allo sfinimento la Nazione giustificandovi con quello che ho sentito dire da un collega della Lega poco fa, tornando di nuovo sul tema superbonus? Provate voi a portare oltre un milione di lavoratori nei cantieri Provate voi a rilanciare l'economia nazionale. Vediamo qual è il vostro coraggio. Oltre alle chiacchiere, portate i fatti.

per il tramite delle Assemblee deputate a rappresentare il popolo italiano, cioè le rispettive Camere che voi mortificate da mesi, a settimane alterne, bastonando una volta la Camera, una volta il Senato... *(Applausi)*. Questo è il luogo della democrazia italiana: non ve lo scordate. scordate. Prima ancora di portare a termine il vostro disegno destabilizzante della democrazia italiana con il premierato, pensateci. Per ora quella italiana è una Repubblica democratica e le Camere hanno voce e la devono avere.

di nuovo cambiato idea: non bastano più i quasi 12 miliardi in spesa corrente, comunque presi dal bilancio dello Stato. Ora state deviando - mi dispiace che se ne sia andato il ministro Fitto - quasi 2,5 miliardi, togliendoli dai fondi per la coesione del Sud, alla Sicilia e alla Calabria? Pensateci. Se non avete idee e risorse, non vi avviate a fare politiche che non potete né garantire né mantenere. Andiamo ai temi di politica internazionale e ai luoghi di guerra. Presidente Meloni, vi sono oltre 18.000 morti a Gaza, di cui 10.000 sono bambini. bambini sono morti nella Striscia di Gaza: un numero che dovrebbe far saltare in aria chiunque, qualsiasi essere umano. Se ognuno di quegli innocenti fosse depositato su questi seggi, ci vorrebbero cinquanta Aule come questa per contenerli. Pensiamoci bene. Oltre 10.000 bambini morti e noi ancora continuiamo a balbettare una posizione non chiara. Diciamo in maniera chiara al mondo non si può utilizzare la scusa dell'attacco criminale di Hamas a Israele per poi fare che cosa? Continuare in un genocidio? Volete portare tutta quell'area a una guerra infinita?

in maniera inequivocabile. Signor Presidente, mi permetto di leggere alcune affermazioni e anche un virgolettato. Cambiamo il fronte e passiamo in Ucraina. All'ultimo G20 un suo omologo ha fatto delle affermazioni almeno nuove, innovative dal suo punto di vista, dicendo che dobbiamo pensare a porre fine a questa tragedia, addirittura il termine guerra e non più operazione speciale. Il suo omologo comincia a fare uno sforzo in quella direzione, mentre noi ci ostiniamo ancora con una politica che ha dimostrato essere fallimentare. Lo stesso suo omologo - non lo nomino, ma è chiaro a chi mi riferisco - ha anche detto che Zelensky non ha mai chiesto di aprire un tavolo e un negoziato di pace; addirittura ha fatto una norma interna, una legge che vieta a chiunque di aprire o proporre tavoli di pace. E noi continuiamo su questa scia? Proviamo a essere i promotori, a metterci capofila della delegazione dell'Unione europea per aprire veramente un negoziato. Quella guerra di logoramento e di sfinimento, oltre a portare migliaia di morti, sta affossando anche le Nazioni dell'Europa, e non solo, per tanti riflessi di natura economica. Non vogliamo vedere solo i profili umanitari visto che qualcuno non li vede. Non è chiaramente solo un problema economico: la vita degli esseri umani

Se sì, con quali atti? Solamente le future forniture o anche quelle con contratti in essere firmati prima? Ci dia delle informazioni chiare, le dia alla Nazione, in modo da poter valutare in maniera attenta qual è la politica che il suo

questi processi di aggressione. Noi invece cosa facciamo? Lei si è astenuta. Come mai si è astenuta su quel voto per l'immediato cessate il fuoco?

l'approccio sulla logica di pacchetto, che lei ha attaccato ferocemente più e più volte ed ora è diventato il suo cavallo di battaglia. *(Applausi)*. Quella logica di pacchetto che ha tanto denigrato ora lei la usa per difendere una posizione scomoda anche nei confronti dei suoi alleati, che chiaramente si sono sempre

abbiamo apprezzato molto il suo intervento di ieri alla Camera: un intervento costruttivo e pragmatico, che dimostra apertura di idee. Basta leggere quello che ha scritto e, se i colleghi lo leggessero meglio, capirebbero che c'è una grande apertura di idee. C'è voglia di approcciarsi all'Europa con il progetto di creare rapporti e non subirli. Per noi ciò è fondamentale perché - a nostro avviso - l'Italia deve sempre andare a testa alta in Europa. di ragionare di numeri e bilanci e di non subire *diktat*, di far capire la posizione dell'Italia sui vari *dossier* e di non subire il compitino a casa da parte di chi in Europa ha sempre fatto la parte del padrone. E purtroppo, negli ultimi anni, abbiamo spesso spesso subito chi guardava l'Italia con sorrisini, chi guardava l'Italia come l'ultima della classe e chi guardava l'Italia come quella a cui far fare il compitino a casa, per poi rimandarci indietro dicendo "tornate un'altra volta". Presidente, è il risultato di un sano dibattito tra le sensibilità dei vari partiti della coalizione, perché è una coalizione fatta da partiti diversi, con sensibilità diverse, ma che hanno la forza di sedersi attorno a un tavolo, confrontarsi e arrivare a una sintesi, grazie al confronto che questo Governo ha con le parti sociali, Presidente. Ieri eravamo a Confagricoltura e il presidente Giansanti, in modo autorevole, ha spiegato ancora una volta qual è la posizione dell'agricoltura italiana in Italia e qual è la posizione da tenere in Europa. E abbiamo preso appunti. È anche sintomo di un processo di ascolto di chi in questo momento è all'opposizione, la cui voce, Presidente, non può restare inascoltata. Questo Governo ha il pregio, contrariamente ai precedenti, di ascoltare chi è all'opposizione, di non deriderlo e di portare in Europa anche idee diverse dalle nostre. Anche l'opposizione rappresenta quegli italiani che non ci hanno votati, ma che comunque ci guardano e che noi stiamo governando. Presidente, i tanti, troppi punti che tratterete denotano, però, anche l'importanza di una revisione del funzionamento di questa Europa: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Commissione europea; tre consessi autorevoli dove la mediazione, spinta da interessi spesso contrastanti, porta a prendere provvedimenti non in linea con le reali necessità dei cittadini europei;

decisioni come quella presa sul quadro economico finanziario pluriennale, dove gli stanziamenti decisi dalla Commissione in tema di immigrazione sono stati quasi azzerati dal Consiglio. Sulla partita dell'immigrazione, Presidente, noi le chiediamo di andare ancora una volta a testa alta - glielo dirò anche dopo - e di spiegare la posizione non solo dell'Italia, ma di tutti quei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che hanno bisogno di di un Paese autorevole come l'Italia che li aiuti. Penso alla Grecia, penso alla Spagna, penso in parte anche alla Francia, al Sud della Francia, penso a Malta, penso a Cipro, penso a quei penso a quei Paesi che hanno bisogno di un capofila che vada in Europa e spieghi ai Paesi del Nord Europa cosa sta succedendo nel Mediterraneo. Questa Europa, Presidente, deve cambiare passo. Questa Europa non può essere lasciata nelle mani dei burocrati, che quasi quasi non sanno nemmeno dov'è l'Italia. E glielo dice un senatore che, quando è andato da Ministro in Europa, in quei quattordici mesi, ha notato che molto spesso ci guardavano e ci chiedevano quasi quasi dove eravamo.

la presidente von der Leyen si ricordi che esiste l'Europa, perché ricordiamo alla presidente von der Leyen che, durante il suo primo intervento al Parlamento europeo (cinque anni fa), la parola "agricoltura" non l'ha nominata neanche una volta. Velocemente, Presidente, alcuni punti che tratterete. Sull'Ucraina siamo a un punto in cui l'Europa si deve proporre come interlocutore di pace. Abbiamo la guerra in casa, contrariamente ad altri, che continuano a indicarci cosa dobbiamo fare. In Europa abbiamo la guerra in casa e non possiamo continuare in questo modo. La nostra proposta, la nostra idea consiste in un piano di pace europeo che veda l'Italia come protagonista. Sul Medio Oriente, Presidente, l'attacco a Israele da parte di Hamas è l'attacco del terrorismo islamico contro la democrazia. Lo statuto di Hamas prevede la distruzione dello Stato di Israele. Questa non è una guerra tra Israele e Palestina, come dice qualcuno, come dicono quelli che vanno in piazza con le bandiere della Palestina e ci raccontano cose che non esistono. Questa è una guerra

dalla parte di Israele, perché vuol dire stare dalla parte della democrazia. Soprattutto, Presidente (e so che tocco anche le sue corde), dobbiamo stare

Sull'allargamento bene, ma attenti a chi ci portiamo in casa, attenti a chi portiamo in Europa. Oggi un bell'articolo sul «Corriere della Sera» ci dice che va bene l'allargamento, ma in modo graduale. Non dobbiamo fare gli errori che sono stati commessi nel passato. Sull'immigrazione, Presidente, una vecchia canzone recitava: «Parole, parole, parole». Non sono le sue, ovviamente. In questi anni - e io da dieci anni sono seduto sempre in questo posto ho sentito solo tante belle parole da parte dei nostri *partner* europei, però i fatti sono altri. Ci hanno lasciati soli a gestire la partita dell'immigrazione. Ancora una volta, Presidente, ci hanno lasciati soli. Ci hanno lasciati soli per poi criticarci quando provavamo a fare qualcosa, quando proviamo a far qualcosa. Quindi, ancora una volta, la esortiamo a difendere i confini del nostro Paese, perché difendere i confini del nostro Paese vuol dire difendere i confini dell'Europa. Infine, mi rivolgo a lei, Presidente, e termino. Parlano degli amici, i colleghi della minoranza; ma chi sono i loro amici?

Siamo all'ammucchiata in Europa e noi a questa ammucchiata, Presidente, non ci stiamo. Questa è l'ammucchiata del "cambiamo tutto per non cambiare niente". Il vostro amico, il premier slovacco, ha fatto leggi durissime contro gli immigrati, sia i clandestini che i richiedenti asilo: begli amici che avete! E poi parlate dei nostri. finestra") *(PD-IDP)*. Signor Presidente, sono molto contento che il senatore Centinaio abbia richiamato un'attenzione verso l'opposizione. Devo dire, senatore, che purtroppo questa notte lei è stato smentito dai fatti.

e tre subemendamenti dei relatori agli emendamenti del Governo. Stiamo lavorando in condizioni che non rispettano né le prerogative dell'opposizione, né quelle della maggioranza.

se avesse lasciato l'Ucraina sola di fronte a questa invasione e che, dopo l'Ucraina, sarebbe stata la volta di altri Paesi e sarebbe iniziato un percorso di instabilità geopolitica europea e, in generale, del mondo occidentale. Su questa posizione, quindi, lei avrà il pieno sostegno dell'opposizione. Lei può parlare tranquillamente a nome dell'opposizione. Questa era la nostra posizione, è stato ricordato qui il treno, ma al di là dei treni e delle fotografie, la sostanza è questa. Lei ha detto una cosa importante ieri, che ho letto dal testo delle sue ha detto che l'Ucraina ha già vinto e sono d'accordissimo con lei. L'Ucraina - e il popolo ucraino - con la sua tenacia e la sua resistenza ha già vinto e lo zar è già stato sconfitto, perché pensava di annettersi gran parte del territorio e non è riuscito a farlo. Purtroppo dobbiamo dire che, se questa è la situazione, se siamo convinti che in fondo non ci sia più alcuna possibilità per la Russia di

aprano dei colloqui per una pace giusta, basata sul rispetto del diritto internazionale. È di questo protagonismo che noi vediamo una certa latenza, sia europea che italiana. Serve questo protagonismo nell'avvio di un tavolo negoziale, perché è il modo migliore per riconoscere la resistenza ucraina, per non fiaccare ulteriormente la popolazione civile ed evitare inutili sofferenze anche al popolo russo, che - così come il popolo palestinese non è responsabile dei crimini di Hamas - non può pagare fino in fondo la volontà di potenza e di egemonia di un'autocrazia che la governa. In questa direzione, invitiamo il Governo ad intraprendere un'azione diplomatica più efficace, costante e più attenta a promuovere delle iniziative che impongano un cessate il fuoco, proprio perché vogliamo la fine delle sofferenze e che da quel cessate il fuoco partano le trattative per ristabilire l'ordine internazionale e i confini, come dice anche il piano di pace cinese. Quindi, sull'Ucraina sull'Ucraina siamo assolutamente convinti che la posizione del Governo, che lei ha espresso, sia giusta. Lei ha detto che dobbiamo pensare che l'Ucraina già vinto, ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo della pace: d'accordissimo. Vorremmo sapere quali iniziative concrete stiamo facendo in questa direzione, perché per una pace giusta e duratura c'è anche bisogno di intraprendere qualche iniziativa concreta. L'altro argomento che è stato affrontato è relativo è relativo alla tragedia mediorientale. È stato detto già dai miei colleghi: viviamo in tempi molto difficili, direi tragici; ben due guerre sono alle porte dell'Europa.

mortale per le democrazie occidentali: la trappola dell'odio. Infatti, da un lato Hamas è riuscito a stimolare un'ondata di antisemitismo in Europa e l'antisemitismo - come diceva Giorgio La Pira - è una malapianta che cresce nell'Occidente, anche cristiano; dall'altro lato, ha provocato e sta provocando un'isteria islamofobica verso i Paesi arabi e i Paesi islamici, come se diritti del popolo palestinese dovesse essere una prerogativa dei Paesi arabi. I diritti del popolo palestinese sono una prerogativa di tutti coloro che credono nei diritti internazionali dei popoli, nei diritti umani e nella dichiarazione universale dei diritti umani. Questo è il punto: noi siamo - e la posizione italiana da questo punto di vista è in perfetta continuità, ancora una volta, con le posizioni precedenti - per i "due popoli, due Stati". Ancora una volta qui però noto una mancanza di coraggio, mi perdoni, perché l'amministrazione americana dice espressamente - e noi lo ribadiamo nella nostra

cominci a mettere in campo delle azioni di deterrenza a questa continua autorizzazione che il Governo israeliano concede sugli insediamenti. È chiaro che tutto questo ragionamento fa parte del diritto internazionale e della coerenza rispetto a una linea di politica internazionale in cui vi sono due popoli e due Stati. Signora Presidente Signora Presidente del Consiglio, non è possibile pensare di ragionare in termini di due popoli e due Stati senza ristabilire il diritto internazionale: non è possibile farlo con l'Ucraina, non è possibile farlo neanche con la Palestina.

Il problema non è quindi essere distanti e mettere a posto le virgole, per così dire, ma avere un'equivicinanza ai due popoli, come ha detto giustamente il Santo Padre.

il problema non è il se, ma il come, signora Presidente: al quinto decreto-legge sull'immigrazione continuate a dire che

gli accordi con l'Albania, secondo noi, sono fallimentari, perché sono fuori dal diritto internazionale e non risolveranno alcun problema.

ma dentro un quadro europeo: questo è il punto fondamentale, cioè il modo. Pensiamo che queste politiche dell'immigrazione non siano né sufficienti né capaci di dare una vera svolta e un vero impulso anche a politiche europee sull'immigrazione. Su questo dovete interrogarvi.

Come avrà notato, le ho dato due minuti in più, perché le ho lasciato concludere un discorso molto, molto lineare,

Presidente del Consiglio, c'è davvero tanta Italia in questo Consiglio europeo, o meglio, c'è tanta azione di Governo italiana nei punti all'ordine del giorno che il Consiglio tratterà a Bruxelles domani e dopodomani. C'è l'Ucraina, che ha visto la posizione italiana chiara e netta da sempre, che ha convinto anche alleati più timidi e oggi forse più stanchi, perché abbiamo sempre detto che per trovare la pace basterebbe che la Russia smettesse di combattere; se invece a smettere di combattere fosse l'Ucraina, non esisterebbe più l'Ucraina e il mondo e la nostra civiltà si dovrebbero arrendere alla legge del più forte. Se oggi l'Ucraina esiste è perché il suo popolo coraggioso non si è arreso all'invasore e perché il mondo occidentale lo ha sostenuto e in Aule come queste e nei Parlamenti del mondo occidentale quasi tutti hanno avuto la possibilità e l'occasione di non andare verso un'astratta pace, ma si sono voluti inviare armi e aiuti perché quella pace potesse esistere davvero, speriamo il prima possibile. È il Consiglio europeo che ovviamente si deve occupare dell'allargamento ad Est dell'attenzione verso l'Ucraina, ma non può dimenticare il Sud e il Mediterraneo. Intanto perché abbiamo a che fare con quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove il Consiglio europeo deve dire a chiare note che Hamas è un'organizzazione terroristica, che Israele ha diritto ad esistere e a difendersi e che in molte di quelle manifestazioni che stiamo vedendo anche in questi giorni teoricamente *pro* Palestina stanno in maniera preoccupante preoccupante riaffiorando sentimenti di antisemitismo e anche, forse, una sorta di collateralismo con chi ha attaccato Israele; è come quando si invitano nelle università terroristi palestinesi a parlare o come quando docenti universitari di tante università italiane fanno ignobili documenti per chiedere di interrompere le collaborazioni tra università italiane e università israeliane. Ci si chiede ancora oggi in quest'Aula perché ci siamo astenuti sulla risoluzione delle Nazioni Unite, ma il motivo è molto semplice ed è stato spiegato più volte: in quella risoluzione, malgrado sia stato richiesto, non c'era nessun momento di condanna di Hamas. L'Italia poteva sostenere questo documento? Oggi ce lo chiediamo ancora in quest'Aula, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle? Che cos'è questo? È collateralismo, è alleanza, è copertura di chi ha attaccato Israele? Lo dico perché noi, d'altro canto, ovviamente dobbiamo sostenere il più possibile l'Autorità nazionale palestinese, che è l'unico vero interlocutore di Israele, del mondo occidentale e dell'Europa. Ma dobbiamo occuparci del Sud del mondo, dell'Europa e del Mediterraneo in questo Consiglio europeo, perché anche il tema dell'immigrazione è un tema che non possiamo più dimenticare, dedicandogli un fondo apposito, sviluppando politiche adeguate, incentivando gli accordi con i Paesi africani. Presidente, lei qualche giorno fa ha detto in un'intervista che possiamo approvare tutte le risoluzioni più belle del mondo, possiamo inventarci tutte le leggi che vogliamo, ma le cose non cambieranno mai se non cambia un atteggiamento, una sensibilità. Lei ha parlato di fiducia reciproca, di capacità di riscoprirsi comunità, di sentirsi parte di un progetto più grande e più alto, un sentimento che in passato ha reso l'Italia ciò che è oggi e che dobbiamo saper recuperare. di quella fame d'Italia, di quella voglia di Italia che giustamente c'è nel mondo e di quanto nel mondo aspettano questa Italia diversa che cominciano a conoscere. È la nostra storia che è stata segnata da questo sentimento che lei ha descritto e che oggi noi tentiamo di recuperare. È l'Italia che fonda la prima università nel mondo come luogo libero per l'insegnamento e dove poter formare i giovani a prescindere dalla nobiltà di nascita. È l'Italia che con navi e con mezzi anche stranieri scopre nuovi mondi e nuove terre. È l'Italia che, già Nazione ma non ancora Stato, per cento di superficie della terra realizza il 70 per cento del patrimonio artistico mondiale. *(Applausi)*. È l'Italia che con i propri missionari mette insieme mondi e Continenti sconosciuti. È la storia di padre Mattei che, partito

Per molti l'Europa nasce qui, grazie a un italiano che ha saputo per la prima volta disegnare un'entità sovranazionale. È l'Italia che tra Stato e mercato dà vita a una terza via della sussidiarietà, del terzo settore, del volontariato, che nella nostra Nazione diventa riferimento per tutto il mondo, che non è solo raccolta fondi o beneficenza, ma sono donne e uomini che diventano angeli del fango, che intervengano negli scenari di crisi, che si donano disinteressatamente e che diventano un modello da copiare. È l'Italia dei nostri giovani in divisa, che difendono, sì, la pace, ma che diventano anche capaci di costruire ponti, ospedali, scuole, contatti e rapporti veri. È questa Italia che abbiamo voglia di recuperare con questo Governo e che vogliamo portare in Europa. È l'Italia che si siede insieme ai tanti Paesi africani per disegnare uno scenario di sviluppo, senza sfruttamento e senza superiorità ed è difficile capire e pensare che sia un progetto vuoto questo del "Piano Mattei", quando i principali *leader* africani sono contenti, accorrono e cercano di costruire insieme a noi questo piano. È difficile davvero dire che non c'è nulla. È l'Italia che si siede insieme ai Paesi arabi per segnare una strada per la pace in Medio Oriente, senza infingimenti e collaborando con tutti. È l'Italia che chiede

che fa l'accordo con l'Albania per dare una risposta sull'immigrazione senza respingimenti o abbandoni in mare, ma senza neanche aperture indiscriminate. È l'Italia che, anche se non è all'ordine del giorno del Consiglio europeo, parla, tratta, spiega e convince sul Patto di stabilità; racconta le sue ragioni, perché vuole vuole il rispetto delle regole, anche senza sconti; non possono, però, esserci regole che si fanno sulla pelle dei popoli, delle Nazioni, delle imprese e dei territori, degli enti locali. Soprattutto, poi, sono regole

A volte si cita Orban, che - lo ricordo sommessamente a tutti - è un Presidente eletto dal popolo ungherese, quindi quando lo si attacca si sta dicendo che il popolo ungherese ha scelto in modo antidemocratico e in maniera addirittura razzista. Vorrei però parlare del *premier* Sanchez, che decide di fare un Governo con gli indipendentisti e i separatisti e per farlo concede loro le immunità, andando contro quello che la Costituzione spagnola prevede *(Applausi)* e contro quello che la stessa magistratura spagnola ha previsto, tant'è che la Commissione europea ha inviato una lettera per chiedere a Sanchez dei chiarimenti. Va bene tutto quando chi governa è di sinistra?

molto interessante e che offre diversi spunti. Come sempre non tornerò su questioni sulle quali ritengo di aver già ampiamente spiegato la posizione del Governo italiano, ma cercherò di rispondere ad alcune cose che mi sono state chieste e di parlare di quelle sulle quali non sono d'accordo.

mutato e per risolvere alcune criticità presenti nei piani che erano stati adottati dai precedenti Governi veniva considerata un'ipotesi impossibile o veniva addirittura derubricata, come ricordavo ieri alla Camera, a una scelta folle che ci avrebbe fatto perdere le risorse del PNRR, portando quasi l'Italia fuori dall'Europa, in questo racconto sempre francamente un po' distorto e distruttivo che non fa stato del ruolo dell'Italia, che non fa stato di quello che noi possiamo ottenere con un po' di pragmatismo e un po' di buon senso. *(Applausi)*. Quello che noi abbiamo dimostrato è che le cose, se fatte bene, si possono ottenere, nonostante il fatto che - sono d'accordo con chi lo ricordava - si è tifato più perché all'Italia non venisse pagata la terza rata del PNRR che alla finale di Coppa Davis. Nonostante questo noi siamo riusciti a ottenere il pagamento della terza rata del PNRR, a essere la prima Nazione d'Europa alla quale viene pagata la quarta rata del PNRR. *(Applausi)*. Ed entro la fine di quest'anno consegneremo tutti gli obiettivi della quinta rata del PNRR e, nel contempo, abbiamo revisionato il Piano per liberare delle risorse e spenderle su priorità che, secondo noi, sono molto importanti. Abbiamo liberato 12 miliardi di euro che abbiamo concentrato sul sistema produttivo italiano, particolarmente sul suo efficientamento energetico. Abbiamo liberato 5 miliardi di euro da investire nelle infrastrutture, in particolare in quelle energetiche, perché - sì, signori - abbiamo una strategia; capisco che possa essere una novità, ma abbiamo una strategia che si lega anche con il tema del Piano Mattei. Collega Delrio, capisco che possa possa dare fastidio che l'Italia finalmente abbia una strategia di politica estera che è anche quella di lavorare per fare dell'Italia un *hub* energetico di approvvigionamento per l'Europa intera, rafforzando le reti e le infrastrutture energetiche, rafforzando la nostra cooperazione internazionale e la diversificazione. Ci abbiamo lavorato anche con lo strumento del PNRR ed è esattamente quello che avevamo promesso che avremmo fatto. Abbiamo liberato le risorse sul diritto allo studio; abbiamo liberato risorse per aiutare l'Emilia Romagna; abbiamo liberato risorse per rafforzare ancora di più il finanziamento sulla sanità e non devo ricordare ancora una volta, al di là di quello che si ripete come un mantra con un piccolo *escamotage* tecnico,

Vi spiego qual è il piccolo *escamotage* tecnico che vi consente di provare a raccontare una storia diversa, cioè di provare a dire che non è vero che oggi sul fondo sanitario ci sono circa 10 miliardi in più di quanti ce ne fossero quando al Governo c'eravate voi, durante gli anni del Covid, nonostante 180 miliardi di euro spesi a debito. *(Applausi)*. La ragione per la quale si fa sempre riferimento al rapporto

Come dicevo, sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare sul PNRR, che dimostra quanto certa propaganda purtroppo poi si scontri con la realtà.

accomodi, senza disturbare. Non si interrompe il Presidente del Consiglio, come qualunque altro senatore, mentre interviene, come ha fatto la senatrice Pirro.

è quello che farò, ma consentitemi di dire quello che penso. Passando al tema del Patto di stabilità, chiaramente questa è materia molto complessa, è stata citata da molti interventi e ho sentito dire anche molte cose Come ho affermato ieri e ribadisco anche in quest'Aula, la trattativa è chiaramente molto serrata e le posizioni di partenza sono molto distanti. Penso che qualche spiraglio si veda e che la posizione italiana - l'ho detto e lo ribadisco - si debba decidere alla fine

anche di difesa dell'Europa. Non avrebbe senso - sono d'accordo con quello ho sentito dire anche dal presidente Monti - che l'Europa, nel momento in cui deve definire la *governance* non tenga conto di ciò che ha incentivato gli Stati nazionali a fare. Noi siamo stati incentivati, anche con il PNRR (che oggi, sul piano dei debiti da restituire, più un peso; poi ne vedremo i risultati quando sarà stato interamente messo a terra), a fare una serie di investimenti su alcune materie e, secondo me, riconoscere il valore di quegli investimenti nella riforma del Patto di stabilità e crescita non serve solamente all'Italia, all'Italia, ma all'Europa intera. Altrimenti si continuano a fare delle cose totalmente miopi; da una parte, si incentivano gli investimenti e, dall'altra, si colpiscono le Nazioni che fanno quegli investimenti sulle regole della *governance*. È una posizione di buon senso. È una posizione pragmatica quella che stiamo portando avanti, sulla quale, come dicevo ieri, siamo ancora lontani, non siamo ancora ad un accordo definitivo, ma non posso non esprimere una punta di soddisfazione per qualche passo avanti che viene fatto. Secondo l'ultima bozza di accordo sulla traiettoria di aggiustamento del rapporto *deficit*-PIL si dovrà tenere conto nel triennio 2025-2027 degli interessi che sono stati maturati sul debito contratto per gli investimenti effettuati in questi settori. punto di partenza; chiaramente la richiesta che continuiamo a fare noi è che ciò non avvenga solamente per questi tre anni. Le posizioni però di altri Paesi sono distanti e, quindi, bisogna capire alla fine dove è che si riesce a raggiungere una sintesi e fare una valutazione serena su cosa sia più utile per l'Italia. Con riferimento a quello che il presidente Monti ha detto relativamente all'apposizione di un veto da parte italiana, io non escludo nessuna

le diverse ipotesi in campo. Io farò tutto quello che posso per far ragionare e per confrontarmi con i miei omologhi sul fatto che quello che stiamo proponendo è utile non solamente a noi. È utile a una strategia. Anche qui,

diversi esponenti della sinistra, del Partito Democratico particolarmente, sui rapporti in Europa, sui compagni di viaggio, sul "con chi si sta e con chi non si sta", se io volessi seguire il ragionamento secondo il quale non bisogna parlare con chi ha posizioni distanti da noi su vari temi, non dovrei parlare nemmeno con la Germania. Nel senso che sul Patto di stabilità la Nazione che ha la posizione più distante da noi non è mica l'Ungheria di Orban, è la Germania di Scholz. Ma è legittimo. È legittimo perché ogni Stato membro cerca di portare a casa quello che ritiene essere meglio per sé o migliore dal suo punto di vista. Purtroppo, signori, accade su ogni *dossier*, con delle maggioranze che sono totalmente variabili. continuo cioè a ritenere che sia un enorme errore in politica estera sovrapporre il rapporto tra Governi alle logiche di partito. È una stupidaggine, consentitemelo, che tra l'altro comporta anche delle enormi contraddizioni. Ricordo una sinistra che mi ha sempre parlato di un'Europa di serie A e di un'Europa di serie B, dove l'Europa di serie B erano per esempio i Paesi di Visegrád. Ma oggi che invece la Polonia è governata da Donald Tusk, continuerete a parlare della Polonia come di una Nazione di serie B o la Polonia magicamente diventerà una Nazione di serie A? *(Applausi)*. La politica estera non si fa così, perché si colpiscono gli interessi della propria Nazione. La politica estera deve saper parlare con tutti ed è quello che cerco di fare io ogni giorno, ben sapendo che su ogni *dossier* - come dicevo - le mie posizioni non si sovrappongono a quelle degli altri, quasi mai, non a quelle di tutti gli altri. E io continuo a rivendicare che è molto più forte in politica estera chi riesce a dialogare con tutti. Se oggi c'è la possibilità di raggiungere degli obiettivi su materie che sono distanti è anche grazie a una posizione italiana e a un ruolo italiano, di una Nazione che è in grado di dialogare con tutti. Questo ci dà una nostra soggettività. Quello che dicevo ieri relativamente alla foto è lungi dall'essere un attacco a Mario Draghi, come è stato letto; tutti sanno cosa penso, particolarmente, della fermezza che Mario Draghi ha avuto sulla questione ucraina, con una maggioranza che era molto difficile da gestire da questo punto di vista. Mi pare che ve lo ricordiate bene. *(Applausi)*. Quello che io cercavo di spiegare è che, proprio perché ho rispetto di quella fermezza, secondo me il il lavoro che è stato fatto e la fermezza che è stata dimostrata non si risolvono nella foto sul treno con i francesi e i tedeschi. Mi dispiace che anche su questo si cerchi di ribaltare il quadro. quel treno l'ho preso anche io, le è sfuggito? Io sono salita sullo stesso treno per andare a Kiev, quindi si figuri se non capisco il valore che questo ha. Però lo dicevo per raccontare che, dal mio punto di vista (è l'impressione che ho avuto stando un anno in Consiglio europeo), c'è stata un'Italia che in passato ha ritenuto che tutto il suo ruolo dovesse essere quello di aspettare e di vedere che cosa facevano Francia e Germania, per poi accodarsi sperando di infilarsi dentro una fotografia. *(Applausi)*. Io non penso che questa sia la politica estera; ma questo non vuol dire che che non abbia buoni rapporti con la Francia e con la Germania e che non abbia le mie foto con Orban, con Scholz, con Macron e con chiunque. *(Applausi)*. Io penso che la politica estera sia

Se avete argomenti, risponderete in replica. Io non è che mi metto a gridare mentre parlate. Dopodiché, non lo vedo solo io che c'è questa differenza. Immagino che voi chiaramente direte "oh, non è vero", ma lo vedono anche molti colleghi europei, che lo dicono e me lo dicono:

C'è uno di questi *leader*, al quale è stata chiesta un'intervista da un quotidiano non esattamente mio amico e che in quell'intervista ha detto questo. L'intervista non è stata pubblicata. ciò non vuol dire che le persone non vedano che oggi c'è un'Italia aperta e pragmatica, che ha il suo punto di vista, che ha una sua soggettività che non si limita a ritenere che, prendendo un caffè con altri due *leader*, si sia risolto il problema e che per questo è forse più rispettata di quanto lo fosse in passato. *(Applausi)*. E che per questo riesce anche a portare a casa qualcosa di quelli che sono i suoi interessi. Dopodiché, collega Monti, sull'allargamento sono molto d'accordo sull'allargamento sono molto d'accordo sul fatto che sia una scelta strategica storica per noi e che bisogna fare tutto quello che possiamo. Chiaramente ho detto, nella mia relazione di ieri, che l'allargamento, particolarmente se immaginassimo domani un'Unione europea con più di

il percorso di riforme che saremo chiamati a intraprendere. Bisognerà lavorare per aggiornare il funzionamento delle politiche: penso alla politica agricola comune, alla politica di coesione; sarà altresì necessario ragionare sul bilancio, sulle modalità di finanziamento delle politiche, sull'efficacia dei processi decisionali. penso che non dobbiamo fare l'errore di partire dal processo decisionale, altrimenti non arriveremmo mai a una soluzione; io penso che dobbiamo partire da ciò di cui si deve occupare l'Unione europea. In particolare, un'Unione europea che domani dovesse contare 32 membri credo che dovrebbe occuparsi di minori materie e di materie sulle quali gli Stati nazionali non competono da soli. Se noi pensiamo che un'Europa a 32 Stati, domani, possa occuparsi di ogni singolo aspetto della regolazione della vita dei cittadini, non andiamo da nessuna parte. andiamo da nessuna parte. La prima cosa da fare - e adesso è il momento, anche se io l'avrei fatto già in passato, ma oggi, secondo me, non si può scappare - è concentrare le competenze dell'Unione sulle materie sulle quali gli Stati nazionali non sono in grado di competere da soli e lasciare alla competenza degli Stati nazionali le materie più prossime

la posizione che l'Italia sta portando avanti, che io ho portato in tutta questa discussione e che continuerò a portare avanti. Credo infatti che sia questo il ruolo dell'Unione europea. Occorre trasformarla finalmente da un gigante burocratico a un gigante politico. Se noi riusciamo ad affrontare questa sfida, dobbiamo avere tutt'altro che paura di avere molti altri Stati membri all'interno dell'Unione europea. Io che non considero l'Unione europea un *club*, come fanno altri (serie A, serie B, serie C, serie D), D), penso semplicemente che non siamo noi che decidiamo chi sia europeo e chi no. Io penso che non dobbiamo chiamarlo allargamento, ma riunificazione. Penso che chi sia europeo lo abbia già deciso la storia e che lo decida la civiltà della quale questi Paesi, dai Balcani occidentali fino all'Ucraina, sono stati e sono portatori. Credo davvero che si debba fare uno sforzo importante, particolarmente in questa fase, per lavorare sul tema di questa riunificazione. Senatore Monti, le posso solo assicurare che, come sempre, noi rispondiamo solo ed esclusivamente all'interesse nazionale italiano, con tutte le iniziative che portiamo avanti. Spero veramente che non tutti gli italiani siano smemorati. In ogni caso, a beneficio di chi dovesse dimenticare, farò sempre la mia parte per ricordare le politiche disastrose di alcuni Governi precedenti, alle quali oggi noi siamo chiamati a porre riparo. Arrivo al collega Lorefice, che mi ha fornito molti spunti, come sempre. Il collega Lorefice accusa il Governo di portare avanti una politica di austerità. Ho già risposto ieri a un suo collega; non so cosa lei intenda esattamente

che sottrae circa 20 miliardi di euro l'anno alla spesa pubblica, risorse che avrebbero potuto essere spese per la sanità, per le pensioni, per i trasporti pubblici e che invece sono state utilizzate per efficientare meno del 4 per cento del patrimonio immobiliare italiano, in gran parte seconde e terze case, mentre più del 30 per cento di queste risorse pubbliche sono finite a banche e intermediari finanziari, contribuendo alla realizzazione di profitti *record*. *(Applausi)*. Per non parlare delle frodi per miliardi di euro che ogni giorno vengono scoperte e penso che qualcuno prima o poi dovrà fare i conti con la propria coscienza per avere immaginato così male *(Applausi)*, che pure nasceva da un intento condivisibile, tanto da trasformarlo nel più grande regalo mai fatto dallo Stato italiano a truffatori e organizzazioni criminali *(Applausi)*, lasciando invece migliaia di aziende e di famiglie perbene in un mare di guai, questione che ora noi cerchiamo di risolvere. Dopodiché, il collega Lorefice rivendica la grandezza dei dati a doppia cifra sul PIL durante il Governo Conte, ma omette un particolare e cioè quello che è accaduto mentre si usciva dalla pandemia con il Governo Conte, che si chiama - c'è un termine economico per definirlo - *dead cat bounce*

La ragione per la quale, a un certo punto, con Conte il PIL è arrivato a doppia cifra è che nell'anno precedente era sprofondato più di quanto fossero sprofondati i PIL di tutto il resto d'Europa *(Applausi)*. Non è una cosa della quale francamente mi vanterei. il collega Lorefice per aver citato i dati Istat, perché questi sono i tre titoli

tasso di disoccupazione cala al 7,6 per cento»; «Istat, nel terzo trimestre + 480.000 occupati su anno». Grazie per averlo ricordato, sono risultati che ci incoraggiano ad andare avanti e a fare meglio. Sempre il collega Lorefice è intervenuto sul tema del trasferimento delle armi a Israele: noi non stiamo trasferendo armi a Israele. Poi mi chiede se ho bloccato l'invio di armi e commesse precedenti: rispetto a questo volevo sapere se intende le armi che il Governo Conte ha venduto a Israele, visto che il Governo Conte è quello che ha venduto più armi in Israele negli ultimi anni

trovo sensazionale che abbiate voluto tornarci: lei nega che il Governo Conte abbia alla chetichella dato l'assenso alla riforma del trattato

al rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari: «La Signoria vostra è autorizzata a firmare l'accordo, recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità. *F.to* Luigi Di Maio». Questa firma è stata fatta un giorno dopo le dimissioni del Governo Conte. Questa firma è stata fatta quando il Governo Conte era dimissionato, in carica solamente per gli affari correnti, contro il parere del Parlamento, senza dirlo agli italiani, senza metterci la faccia e con il favore delle tenebre. Capisco la vostra difficoltà, capisco il vostro imbarazzo, ma dalla storia non si esce, perché la propaganda si può fare, ma poi rimangono i fogli a dimostrare la serietà di chi parla e questo foglio dimostra la scarsissima serietà di un Governo che, alla chetichella e in silenzio, prima di fare gli scatoloni lasciava questo pacco al Governo successivo.

Son qui da tanto tempo e ho visto applausi più calorosi per questioni almeno altrettanto importanti, mettiamola così.

popolazione civile di Gaza (è una cosa che ci viene riconosciuta anche da tutti i Paesi arabi e islamici): come sapete, abbiamo una nave, la Vulcano, allestita

Gaslini, quando mi sono recata lì per un progetto congiunto con gli Emirati Arabi Uniti per la cura dei civili palestinesi. Come voi sapete, stiamo tentando di capire se ci siano le condizioni minime di sicurezza per allestire un ospedale sul territorio della Striscia di Gaza. Come sapete, anche a livello internazionale continuiamo prevalentemente a dialogare con i Paesi arabi per evitare un'*escalation* regionale di questo conflitto e a passare messaggi di moderazione e di ragionevolezza anche al Governo israeliano. La ragione per la quale ci siamo astenuti è che la mozione era sbilanciata, era sbilanciata, perché, da una parte, proponeva cose condivisibili e, dall'altra, non voleva riconoscere neanche un riferimento ad Hamas e a quello che è accaduto lo scorso 7 ottobre. Penso che un voto diverso avrebbe sbilanciato l'Italia rispetto a una posizione che tutti riconoscono essere di assoluto

so che la proposta di un cessate il fuoco è una di quelle che si portano avanti, però nasconde un'insidia, ce lo dobbiamo dire: dire: oggi un cessate il fuoco in Ucraina equivarrebbe a fotografare la situazione esistente e, in buona sostanza, a dire che diamo per persa una parte del territorio ucraino che è stata occupata e annessa; è quella l'insidia che crea la difficoltà, in assenza di passaggi che invece si cerca di continuare a fare, partendo da un piano di pace proposto dall'Ucraina. Ho sentito dire, sempre ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che la Russia praticamente vuole la pace e l'Ucraina no: l'ho già sentita questa tesi, l'ultima volta l'ha esposta Putin al G20 al quale ho partecipato ed è esattamente quella che la propaganda russa chiede di ripetere evidentemente a chi la segue, ma non è il mio punto di vista.

per portarli su una posizione di mediazione che però deve andare verso una pace giusta, nella quale si riconosca la differenza tra chi è aggredito e chi è aggressore.

si cerchi di fare tutto il possibile per smontare un lavoro faticoso e molto difficile che il Governo sta portando avanti. Mi ha particolarmente colpito la reazione del Partito Democratico sulla vicenda dell'accordo con l'Albania, perché sicuramente non lo si può considerare in violazione del diritto internazionale e questo mi pare sia stato chiarito da tutti, benché ci fossero italiani che correvano dietro a tutti i commissari europei, a tutti i *leader* europei, cercando di portarli a dire che era in violazione del diritto dell'Unione europea *(Applausi)*, ma non ci sono riusciti e quindi mi pare ormai pacifico che l'accordo non viola il diritto internazionale, non viola il diritto nazionale, non viola il diritto europeo. Al di là del fatto che lo si possa condividere o meno, comunque, francamente sono rimasta basita

con i valori della sinistra e quindi non vedo niente di male nel fatto che il *premier* Rama voglia accogliere dei migranti (voi l'avete fatto per una vita e non è che vi abbiano cacciati dal Partito socialista europeo); in secondo luogo, perché penso che tentare di cacciare qualcuno che ha la colpa di aver aiutato l'Italia, che è la Nazione che anche voi rappresentate in quest'Aula, la dica lunga sul punto di vista che si ha rispetto al fatto che si di partito agli interessi complessivi della Nazione. Penso sempre che gli interessi complessivi della Nazione si debbano anteporre a quelli del partito, e non è quello che ho sempre visto da parte della sinistra. *(Applausi.

che illegittimamente occupano il suolo ucraino prima della parte relativa all'immediata cessazione delle operazioni belliche, quindi l'impegno sarebbe ad adoperarsi in sede europea ed internazionale per il ritiro delle Forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino

perché in fondo Draghi non è la Madonna Pellegrina ed è del tutto legittimo che venga attaccato da una rappresentante che era all'opposizione.

qualcosa che è stato inventato in quest'Aula - anche se era da un'altra parte -, nel Senato tanti anni fa e che si chiama *auctoritas*, signora Presidente del Consiglio. L'*auctoritas* è una forza morale, non la forza che deriva da una carica pubblica; non deriva dall'*imperium*, dal fatto di essere Presidente del Consiglio; è una forza che deriva dal prestigio, dal *cursus honorum* fatto, dalla capacità di rivolgersi, come Draghi faceva in quanto Presidente, non alla sua parte, ma a tutta l'Italia, evocando uno spirito repubblicano unificatore.

retti, nel senso di dire le cose come stanno, riconoscendo responsabilità ed anche errori. In questi brevi minuti di intervento, proverò a dire con obiettività quello che condivido e quello non condivido.

la sua linea di politica estera e penso che non sia stato facile mantenerla, soprattutto perché nella maggioranza ha persone che un pochino, soprattutto sull'Ucraina, con i russi hanno avuto a che fare. Dunque bene, avanti così. Lei, Presidente del Consiglio, ha richiamato il fatto che è riuscita a modificare il PNRR in accordo con la Commissione. È vero, e molti di noi, me compreso, pensavano che non fosse possibile. Ho fatto i complimenti al ministro Fitto. E se il ministro Fitto farà, come io spero, un grande piano Industria 4.0 che ci metta al passo con quello che sta facendo la Germania e con quello che fanno gli Stati Uniti, sarà un bene per l'Italia. Dopodiché, signora Presidente del Consiglio, con la stessa nettezza mi permetto di dire che non si tratta di un risultato straordinario. Il risultato straordinario è se riusciamo a spendere i fondi del PNRR. Allo stesso modo mi permetto di farle notare che quella sul MES in quest'Aula è una posizione delirante da parte di tutti: vi state tutti accusando su chi ha mollato prima la contrarietà a una cosa che comunque sappiamo che ratificheremo.

profondamente convinto del fatto che non si possa tollerare l'immigrazione irregolare e che i flussi dell'immigrazione irregolare vadano interrotti. L'accordo con la Tunisia era un inizio su cui bisognava lavorare per farlo funzionare. quell'accordo, da noi è arrivato un apprezzamento, perché non si può fare altro. Non si può pensare di dire al Paese che chiunque vuole venire può farlo, perché è una follia: siamo ai confini dell'Europa. Ma io mi domando come le sia venuto in mente l'accordo con la Tunisia. È una cosa che non è, amici della sinistra, una violazione del diritto internazionale, ma una violazione della razionalità, perché sono pochi migranti su 160.000 arrivati; costa un sacco di soldi e ce li rimandano indietro, se non li rimpatriamo. Mi avvio a concludere. Potrei parlare del Patto di stabilità. Qui c'è un dato che alla fine conta: lei deve parlare a tutto il Paese, soprattutto quando in ballo ci sono questioni che andranno oltre il suo Governo e che saranno più lunghe del suo Governo. Draghi può essere criticato per qualsiasi cosa, è legittimo,

così si sale alle stelle, ha scritto ieri, credo, l'ufficio stampa della manifestazione fondata dal *premier* Meloni, Atreju. Sì, Presidente, è evidente che la sua è un'infinita storia d'amore, se non di condivisione, con il popolo italiano. *Sic itur ad astra* è proprio la strada tracciata da lei, presidente Meloni, nel primo anno del suo Governo, che sta mettendo l'Italia al centro del sistema solare, politico, economico, europeo ed internazionale, rispettata da tutti. *Fact checking* solo sui contenuti del Consiglio di domani. È notizia di ieri che grazie all'accordo del *premier* Meloni con la Tunisia il flusso dei migranti verso i nostri confini sta finalmente diminuendo. Abbiamo incassato per primi - è stato detto - la quarta rata del PNRR e l'Unione europea ha dato il via libera alla modifica dello stesso. Abbiamo tenuto la schiena dritta e la teniamo sulla modifica del Patto di stabilità. Abbiamo dato impulso all'allargamento ai Balcani. L'accordo con l'Albania è stato subito preso ad esempio da Germania, Austria, Francia e Inghilterra. Abbiamo ribadito la ferma collocazione dell'Italia nei valori della NATO e il sostegno incondizionato alla sovranità e al popolo ucraino. Le Borse europee e la Borsa di Milano volano. Tutte queste cose hanno fatto sì che il nostro *premier* sia risultato tra le quattro donne più influenti al mondo e secondo la celebre rivista americana «Politico» addirittura la persona politica più concreta d'Europa. Non è una nostra invenzione, sono gli altri a dirlo. Con questo *background*, che ci rende orgogliosi di essere italiani, il *Premier* si presenta al Consiglio di domani. È per questo che annuncio sin da subito che il Gruppo che presiedo condivide *in toto* la relazione del Presidente del Consiglio e voterà convintamente la risoluzione di maggioranza che dovrebbe essere condivisa, con questi risultati certificati, anche dall'opposizione, che invece si ancora ad una foto. Ribadisco quello che è stato detto già dal *premier* Meloni. L'affondo era nei confronti del Partito Democratico, non certo del *premier* Draghi. Vi posso dire però che non vi fa onore usare l'ex *premier* Draghi come un feticcio, vi manca la bussola, cercatela nelle idee, non nelle persone. Questa nuova riunione del Consiglio europeo dovrà affrontare ancora una volta temi e situazioni che sono terribilmente importanti, drammatiche e non di facile soluzione, ma avrà l'Italia protagonista. Parliamo dei terribili eventi che hanno insanguinato e continuano ad insanguinare il Medio Oriente, l'angoscia profonda per Israele, ma anche per le vittime palestinesi, per gli ostaggi, prede innocenti di una ferocia che solo il fanatismo terroristico e ideologico poteva concepire, obnubilando la ragione e annichilendo il comune senso di umanità. Quella del Medio Oriente è una crisi che drammaticamente ci riguarda tutti direttamente. Il nostro mantra dovrebbe essere che la libertà dell'Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme, perché è volto a minare i valori fondanti dell'Occidente e del diritto internazionale. Ci riguarda direttamente per i temi che sono relativi ai flussi migratori, delle connivenze tra i flussi migratori irregolari e il terrorismo. Noi non possiamo non rinnovare prima di tutto piena solidarietà e pieno sostegno a Israele e al popolo israeliano.

come strumento di difesa, ma le coscienze e le idee che sono sempre state la forza della nostra civiltà. Per questo è necessario che noi ed Israele insieme ci si faccia promotori nei confronti di tutti gli Stati europei, Presidente, affinché tutti insieme si scriva una nuova costituzione europea che abbia come faro le radici giudaico-cristiane, cioè la nostra storia, i nostri valori fondanti e magari si inizi insieme il processo di adesione ad Israele, ponte naturale del nostro continente all'Unione Europea. Combattere l'indifferenza come eredi anche noi di coloro che stanno subendo gli abomini di questo nuovo Olocausto è la nostra battaglia campale perché è nell'indifferenza, cui troppo spesso la nostra società cede, che la cattiveria e la violenza trovano terreno fertile per germogliare. Anche in un'occasione drammatica come questa dobbiamo avere il coraggio e la forza, che a lei sicuramente non fanno difetto, Presidente - di proseguire nel difendere il ruolo fondamentale dell'Italia e dell'Europa in quell'avamposto che è la culla della nostra civiltà e della nostra tradizione e che si chiama Mediterraneo. Proprio per questo occorre continuare a lavorare con la diplomazia, con la politica internazionale, internazionale, con i corridoi umanitari, con gli aiuti di cui l'Italia è capofila, per non cadere in quella che lei ha giustamente definito più volte la trappola dello scontro di civiltà, proseguendo dunque nel dialogo e nelle relazioni bilaterali con i Paesi arabi e musulmani moderati e ragionevoli. Noi, presidente Meloni, siamo dalla parte giusta, quella che si chiama la *right side* (non a caso si dice che è giusto e di destra tutto ciò che è *right*), di chi vuole lavorare insieme per impedire un'*escalation* del conflitto e per arrivare ad una soluzione strutturale sulla base della prospettiva "due popoli, due Stati", prospettiva che deve avere come presupposto, da parte di tutti gli attori presenti nella regione, il riconoscimento all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele. E noi italiani faremo da scudo, affinché nelle piazze italiane, come nelle piazze europee, come nelle piazze dell'Occidente, cessino i rivoltanti rigurgiti antisemiti. Dall'altra parte, Presidente, ci raccomandiamo affinché sostenga, senza se e senza ma, come già sta facendo in Europa, tutti gli aiuti umanitari possibili per i civili inermi della Striscia di Gaza, che subiscono questa guerra senza averla voluta, perché l'attacco di Hamas è un attacco contro i palestinesi pacifisti che vorrebbero vivere tranquillamente e che invece, loro malgrado,

la direttrice del Mediterraneo, che conosciamo e che dobbiamo combattere con il confine esterno dell'Unione, e la direttrice balcanica, di cui poco si parla. Ma i nostri Servizi di *intelligence* continuano ad allertarci e sappiamo che quella è la direttrice attraverso la quale il rischio di infiltrazione islamica è molto più forte ed è quella che dobbiamo controllare. A tal proposito vorrei ringraziare - e non è un ringraziamento retorico - gli uomini e le donne e delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e dei Servizi, per il lavoro che quotidianamente svolgono per prevenire e contrastare tutte le forme di terrorismo e i rischi di infiltrazione, assicurando alla giustizia i fondamentalisti pronti a colpire e garantendo dunque la sicurezza della nostra Repubblica. Viviamo una fase drammatica e la nostra identità liberale, cristiana e democratica rischia di trovarsi in difficoltà e sotto attacco. È per questo che riteniamo non essere più rinviabile la priorità di un allargamento ai Balcani occidentali, che attendono ormai da decenni di poter entrare nell'Unione. È stata molto importante la sua prima visita a Belgrado negli scorsi giorni, così così come la straordinaria accoglienza che le è stata tributata, e la sua indicazione sull'accelerazione del "chi ha tempo non aspetti tempo", riguardo l'accesso dei Balcani occidentali nell'Unione. Questo è un tema che sarà da patrocinare attentamente, combattendo la resistenza di altri Paesi e Stati membri, come per l'Ucraina. Il Consiglio europeo è chiamato inoltre a ribadire, senza se e senza ma, il proprio sostegno all'Ucraina dal punto di vista diplomatico, economico, militare e umanitario. L'Ucraina deve rimanere una priorità nell'agenda europea. Ma l'Italia è chiamata anche, grazie alla sua empatia e capacità di costruire ponti, Presidente, al suo ruolo naturale di portatore di pace. Da un lato vanno intensificati gli sforzi per garantire la protezione umanitaria e l'assistenza civile e militare all'Ucraina per il tempo necessario alla fine delle ostilità, per la ricostruzione del Paese e per determinare condizioni di sicurezza. Dall'altro, bisogna rilanciare lo sforzo economico e diplomatico, per realizzare una formula di pace, per una pace giusta, complessiva e duratura. Nell'ambito della discussione sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sappiamo di avere di fronte partite che non possiamo perdere. Per questo sarà importante sollecitare l'Unione a integrare il bilancio con opportune risorse sul capitolo immigrazione, ma anche e soprattutto sul capitolo costo del denaro, per prevenire una nuova accelerazione dell'inflazione e il rischio di un nuovo *shock* energetico. Sarà indispensabile non perdere di vista un obiettivo: tutelare le famiglie e le imprese, soprattutto quelle maggiormente esposte ai rincari energetici (come abbiamo fatto noi in Italia, ad esempio) e alla stretta creditizia. Sono sfide che vanno affrontate con la giusta dose di coraggio da parte dell'Europa, in cui noi crediamo fortemente. Sulla riforma del Patto di stabilità, infine, noi sosteniamo chiaramente la posizione del suo Governo. Gli investimenti pubblici collegati all'attuazione dei programmi europei devono essere trattati in maniera preferenziale. L'Unione europea dovrà necessariamente trovare un nuovo equilibrio, senza dimenticare però che la crescita è l'elemento più importante per rendere sostenibile il debito. Signor Presidente del Consiglio, infine le affidiamo queste nostre istanze, sapendo che le stiamo mettendo nelle mani di una persona capace, sì, ma soprattutto profondamente innamorata della sua Nazione. La incoraggiamo a proseguire con la massima determinazione, la competenza e la fermezza che la contraddistinguono nella difesa degli interessi legittimi del nostro Paese, in quanto è chiaro a tutti che questi coincidono con un rafforzamento dell'Europa, come sognata dai padri fondatori. Solo un'Italia forte renderà l'Europa il sogno auspicato dai popoli europei. Siamo fieri di lei, Presidente. Grazie.

cose che sono state dette. Il presidente Meloni ha parlato di tifo contro il pagamento della quinta rata del PNRR o di fastidio di qualcuno per il fatto che sia stato fatto il Piano Mattei. Ebbene, io respingo con fermezza l'accusa di avere tifato contro e di aver provato fastidio. Noto che, se di tifo si deve parlare, l'unico tifo che vedo qui è quello che proviene dai banchi di centrodestra, in maniera così entusiasta e appassionata che qualche volta mi viene da pensare che stia per apparire uno striscione con scritto «Forza Meloni». che è vietato dal Regolamento del Senato e che il nostro presidente La Russa vigila in questo senso e lo impedirebbe. Per quanto riguarda la Polonia, signor Presidente, il presidente incaricato Donald Tusk ha dichiarato oggi che la Polonia deve tornare a essere protagonista in Europa, un ruolo che aveva perso col Governo precedente. Lo dice lui e non è certo esponente di un partito di sinistra. Riguardo alla considerazione fatta sull'Europa del futuro, che dovrebbe diventare più federalista - per così dire - accentrando alcuni poteri, ma diventando politicamente rappresentante di una in cui gli Stati si riprendono una serie di competenze, da portare avanti per conto loro, io spero che questa impostazione di pensiero riguardi anche lo Stato italiano rispetto agli enti locali. Sappiamo che, invece, il convincimento di questo Governo, ma in generale della nostra struttura statale, è di accentrare nello Stato e di non delegare. Presidente Presidente Meloni, credo che la Giorgia Meloni che da tempo ormai parla di difesa dell'Ucraina, che usa parole di grande equilibrio sul Medio Oriente, che parla convintamente di allargamento dell'Unione, di un'Europa sempre più integrata attraverso regole condivise, in grado di bilanciare crescita e stabilità, che fa propria l'agenda di Ursula von der Leyen e delle grandi famiglie politiche europeiste, europeiste, non sia neanche lontana parente della Giorgia Meloni degli scorsi anni, quella che usava parole di fuoco contro l'Europa delle banche e dei grigi burocrati di Bruxelles, che sottraevano sovranità agli Stati membri e all'Italia. La presidente Meloni parla di rinnovata credibilità e noi siamo molto felici, se davvero è così. Mi si consenta, però, di dare qualche piccolo suggerimento in merito. In primo luogo, quando si parla di credibilità, si deve pensare non solo alla propria immagine personale, ma anche alla credibilità dell'intero Paese.

E, soprattutto, chi non sarà legittimato a pensare che qualsiasi cosa Giorgetti dica a Bruxelles può essere rinnegata a Roma? Una vera *leadership*, Presidente, valorizza i collaboratori, non li squalifica, soprattutto davanti agli occhi dell'Europa e del mondo. Un altro consiglio: ci eviti le lezioncine sul PNRR e sui migranti. La rinegoziazione del PNRR corrisponde a un chiaro disegno politico di accentrare le risorse e di toglierle dalla mano pubblica dei Comuni e degli enti locali, per metterle in quelle dei grandi gruppi: esattamente il contrario di quello che sarebbe corretto fare dal nostro punto di vista. Il tutto, con l'effetto di ridurre il potenziale di crescita degli investimenti del PNRR, esattamente come certifica l'ultima Nota di aggiornamento al Per quanto riguarda i migranti, quello che è stato fatto in Albania è un accordo costoso e probabilmente inutile, un'ulteriore iniziativa di distrazione di massa, che è la specialità del Governo attuale. È buono soltanto per distogliere dal tavolo il tema dei mancati accordi bilaterali coi Paesi di provenienza, che andrebbero invece fatti. È figlio di una logica vecchia, quella per cui i migranti da gestire sono un problema di ordine pubblico. Sappiamo invece quante aziende hanno bisogno di manodopera e sulla manodopera di cui potranno disporre in futuro è appeso il loro destino. Il terzo consiglio: non confonda i numeri macroeconomici, Presidente, con tanto di elencazione dei giudizi delle agenzie di *rating*, con la condizione reale in cui versa il Paese. Io non elencherò i numeri sul lavoro povero, sulle liste di attesa in sanità e su tutte le altre questioni che il Governo conosce bene. Ma mi limito a citare un altro numero: 200.000 200.000 sono le famiglie che nel 2023 hanno saltato le rate di un mutuo a tasso variabile; 200.000 sono le famiglie che vivono nell'angoscia e che sono la spia di un malessere profondo e di una paura del futuro che attanaglia troppi italiani. Questo, sì, richiederebbe scelte davvero coraggiose: il salario minimo e una forte lotta all'evasione fiscale per recuperare le risorse e mettere in campo vere politiche per la famiglia e la crescita economica. Da ultimo, Presidente: sul 2024, senza ricorrere all'abusata citazione di chi pensa alle prossime elezioni e di chi alle prossime generazioni, ci accontenteremmo che lei sia conseguente fino in fondo. Non mi scandalizzo che forze politiche come quelle dell'attuale maggioranza competano tra loro - è un principio della politica ma mi angoscia pensare che questa competizione si giochi sulla pelle dell'interesse nazionale, magari portando il terzo Paese dell'Unione - siamo noi - a non sostenere il prossimo Presidente della Commissione europea. Mi angoscia pensare a cosa rappresenta quella destra, riunitasi recentemente a Firenze; i bulgari che dicono che l'Europa unita è una minaccia per la civiltà e i portoghesi che propongono di punire le donne che abortiscono,

mi auguro che questo coraggio lei lo trovi, signora Presidente del Consiglio, a partire dal prossimo confronto in Europa. non c'è Italia forte senza un'Europa più forte. Non c'è un'Europa più forte senza un afflato solidaristico e un rilancio del processo di integrazione. Presidente, le faccio i migliori auguri per il prossimo impegno in Europa. la relazione della Presidente è stata una relazione abbastanza normale, non vorrei dire quasi burocratica. Molto più interessanti sono state le repliche, anche quelle che non condividiamo, dove la Presidente del Consiglio ha sfoderato la sua *vis* polemica e *ars* oratoria con indubbia capacità e dalle quali cerchiamo di trarre un po' di considerazioni, augurando comunque alla Presidente in bocca al lupo, perché - lo diceva molto bene Spagnolli in un intervento che condivido dalla A alla Z, a parte la dichiarazione di voto finale noi comunque facciamo il tifo per il nostro Governo e la nostra Presidente quando vanno in Europa. Ci sono almeno cinque punti però, Presidente, che mi lasciano perplesso e sui quali la invitiamo a riflettere per il futuro. Il primo: io ho trovato debole la relazione nella parte in cui non si affronta la vera grande questione che c'è. Da cittadino europeista - direi molto più convinto di altri in quest'Aula - io sono terrorizzato per il futuro dell'Europa. Secondo me, noi stiamo sparendo politicamente - oltre che demograficamente, ma questa è un'altra storia - e non siamo più, purtroppo, sulle mappe della geopolitica. Non Non è certo colpa del Governo italiano, ma nemmeno della Commissione o del Consiglio: è un fatto storico-culturale, dove però bisognerebbe che i nostri *leader* a Bruxelles facessero suonare una campanella o un segnale d'allarme e in questo ci fosse una risposta politica. Faccio un esempio: la presidente Meloni dice giustamente Governo è per l'allargamento e questo viene poi sottolineato negli interventi della maggioranza. L'allargamento ai Balcani è un concetto sacrosanto: chi conosce la storia sa che, se nei Balcani non ci si mette mano, poi succedono problemi. Però, il tema dell'allargamento pone una domanda su che tipo di Europa vogliamo. Noi pensiamo di avere un'opinione diversa dalla sua. Noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa, noi siamo perché l'allargamento produca una Commissione davvero politica. Questo vuol dire superamento del diritto di veto, Europa a più velocità, non retorica dell'Europa delle Nazioni, elezione diretta del Presidente, e non solo del Consiglio, ma anche del Presidente della Commissione. Questa idea di Europa non è uscita nel dibattito degli ultimi giorni. Le auguriamo di potersi fare promotrice di una discussione perché per noi l'Europa, così com'è, finisce. Il secondo punto è il Patto di stabilità. Presidente - mi perdoni

prestito, e un terzo a fondo perduto, e quindi 65 miliardi. Di questi assumiamo che ci sia il 3 per cento di interessi come spesa media e, alla fine, abbiamo un guadagno tra l'1,5 e i 2 miliardi annui, che vuol dire lo 0,1 del PIL.

L'Italia oggi gode del prestigio, secondo la presidente Meloni. Io faccio il tifo per lei - finché c'è lei, poi farò il tifo per un altro e ovviamente lavoro affinché ce ne sia un altro, ma diciamo che, finché c'è lei, faccio il tifo per lei ma non è così. Presidente, la settimana scorsa si è votato perché una cosa è raccontare i titoli dei giornali, altra sono i risultati concreti. C'era da nominare il Presidente della Banca europea per gli investimenti: siamo arrivati terzi su tre; ha vinto la spagnola Calviño, seconda è arrivata la Vestager e terzo Franco.

il rinnovato prestigio del Paese esiste nei vostri film, nei vostri *post* straordinari. Ha detto che non si può fare politica estera con le foto: l'ho pensato anch'io, quando l'ho vista fare la foto con Modi, bellissima. Oggi, per provare a commentare il profilo Instagram della Presidente del Consiglio, bisogna sapere l'hindu: è un'operazione geniale, bellissima, che davvero ammiro e lo dico sinceramente, senza ironia, anche perché deriva da una serie di considerazioni che non possiamo fare su come la propaganda indiana ha raccontato l'utilizzo dei *social*. Bellissimo. Però, Presidente, detto che «Melodi» è affascinante per ragionarne tra di noi, in politica estera lei in questo momento ha le copertine dei giornali, ma non i risultati. E non si permetta, Presidente - lungi da me l'idea di difendere il PD - le battute contro il PD, Edi Rama e il Partito socialista europeo, che ora sono anche simpatiche, per carità di Dio. Ritengo però che sul Patto con l'Albania lei faccia bene a dire che non c'è alcuna violazione di diritti e chi la attacca su quello, come al solito, fa il suo gioco. Il tema è che sul Patto con l'Albania la penso come Edi Rama, che ha detto alla stampa albanese che a loro non cambia niente; a loro non interessa niente; alla Meloni serve, perché deve fare le elezioni. Allora, mettere 70 milioni di euro perché voi dovete fare le elezioni, va bene; insomma, non tanto. Almeno, però, si risparmi di maramaldeggiare sul Partito socialista europeo. È evidente che nel PD ci sono varie correnti - ho un *master* in materia e siamo tutti esperti del settore - ma non può mettere la bocca anche su come funziona il Partito socialista europeo. Pensi ad Abascal, signora Presidente del Consiglio. Pensi ai polacchi, signora Presidente del Consiglio. Non si metta anche nella logica di rissa contro il Partito socialista europeo. Pensi ai suoi alleati, a cui auguro in bocca al lupo, perché ultimamente non gli sta andando benissimo. Finisco

quando c'era il Governo Berlusconi, colei che ora fa la Presidente del Consiglio era Ministro. In quest'Aula, la Presidente del Consiglio è la donna che è stata più giorni al Governo, tranne Dario Franceschini e Maurizio Gasparri, ma *ad impossibilia nemo tenetur*, per superare quei due, per cui va bene. Quindi, la Presidente del Consiglio che si dipinge come *underdog* - e fa benissimo dal punto di vista della sua narrazione - è una Presidente del Consiglio che stava al Governo quando è nato il MES. il MES. Voi avete il diritto di dire di no al MES. Ma, Presidente del Consiglio, faccia votare il Parlamento. Come è possibile che lei, che ci deliziava dei suoi commenti dallo scranno di deputata attaccando il Governo perché non al Parlamento di discutere le leggi di bilancio, ci abbia nascosto la legge di bilancio che arriverà, se ci va bene, il 19 dicembre per la prima volta in Senato e ci abbia nascosto la possibilità di discutere del MES? Votiamo sul MES, colleghi. Uscite dalla retorica per cui siete soltanto una parte della *clac* organizzata. Votate, dividetevi, se qualcuno è per il MES e qualcuno è contro il MES. Venite in Parlamento e vediamo anche le nostre contraddizioni. *(Applausi)*. Io voterò a favore, ma è bello che ci sia un confronto, altrimenti la retorica sulla democrazia parlamentare fa la fine della retorica sul prestigio internazionale e sul Patto di stabilità, e diventa fuffa. Il fatto che lei Il fatto che lei faccia melina sul MES non le fa onore, perché lei è la donna dei "sì sì" e dei "no no". Lei è la donna che ha fatto una carriera su questo. Ma sulla vicenda Draghi - se lo lasci dire, Presidente, premesso che, secondo me le è venuto male il passaggio e succede a tutti, figuriamoci

Quando Mario Draghi ha preso il treno e non si è fermato a Ciampino con una sosta non autorizzata. *(Applausi)*. Quando Mario Draghi ha detto qualcosa in questo Paese, ha portato l'Italia ad avere quell'alta autorevolezza e quel prestigio. Mi auguro per lei, Presidente, che anziché attaccarlo cerchi di copiarlo. Non può che farle bene.

state citate, credo sia giusto cominciare dalle due tragedie in corso ai confini dell'Unione, cioè le guerre a Gaza e in Ucraina. Una intera popolazione, quella di Gaza, è vittima oggi di una punizione collettiva, di una catastrofe umanitaria: milioni di persone sono senza più case, senza servizi sanitari, senza cibo, senza un posto dove ripararsi, costrette a vivere sotto i bombardamenti. E questo avviene mentre in Ucraina la guerra non accenna a finire. La possibilità di risolvere il conflitto con una vittoria militare, colpevolmente perseguita anche dal Governo italiano, si è dimostrata una nefasta chimera. Ora, sulla drammatica vicenda israelo-palestinese, penso che l'Italia dovrebbe davvero provare fino in fondo a spendere il proprio peso. Dovrebbe chiedere la fine dei bombardamenti, il rifornimento di generi di vitale necessità alla popolazione di Gaza, alla protezione dei civili, il rilascio degli ostaggi di Hamas. E soprattutto dovrebbe adoperarsi, Presidente, affinché le richieste delle istituzioni internazionali, a partire dall'ONU, non rimangano lettera morta. lettera morta. Noi crediamo che la soluzione dei due popoli e dei due Stati, nonostante tutte le criticità, nonostante le tante ipocrisie - una per tutte è stata ricordata, gli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania - resti ancora l'unica per mettere fine ad un conflitto che mette a rischio da ogni punto di vista anche noi. Le vorrei dire, Presidente, che riconoscere lo Stato di Palestina è il primo passo urgentissimo e necessario. *(Applausi)*. L'Italia e l'Europa dovrebbero anche prendere atto dell'impossibilità di risolvere la situazione in Ucraina senza la diplomazia, senza una trattativa che potrà esserci soltanto quando tutti accetteranno la realtà. Quella guerra non può e non potrà concludersi con un vincitore e con un vinto. In queste guerre, signor Presidente, c'è un tratto comune sul quale sarebbe utile che tutti riflettessimo: in entrambi i casi prevale e ha prevalso la tentazione di risolvere tutto esclusivamente sul piano della forza, senza diplomazia, senza visione strategica. Quando noi abbiamo provato, molto spesso in solitudine, a sollevare questa esigenza, ci è stato risposto che questo significherebbe darla vinta ai prepotenti, agli invasori, ai terroristi. Io credo che adesso sia il momento di dire che la verità è tutt'altra: la si dà vinta a Putin, la si dà vinta a Hamas, la si dà vinta ai coloni, la si dà vinta ai nazionalisti israeliani quando si accetta il loro terreno, quando ci si muove cioè soltanto sul piano della forza. *(Applausi)*. È esattamente quello che vogliono loro, non certo quello che temono. Inoltre, tra i danni immensi già provocati dalla guerra in Ucraina c'è anche quello sul principale obiettivo strategico che l'Unione si è data, cioè la riconversione ecologica. Quel traguardo rischia di essere derubricato a esigenza secondaria e in questa retromarcia, purtroppo, il Governo italiano è *(Applausi)*. Non passa un giorno, Presidente, senza una vostra dichiarazione che smentisce gli obiettivi del *green deal* europeo. Bisogna invece fare il contrario: tornare al perseguimento della riconversione ecologica non solo a parole, con l'impegno a porre fine entro il 2030 alla sovvenzione per le fonti fossili, per esempio con l'adesione dell'Italia all'alleanza dei Paesi impegnati a non concedere autorizzazioni per l'estrazione dei combustibili fossili e con la rinuncia ad utilizzare il Piano Mattei per sfruttare le fonti fossili dell'Africa. Il suo Governo, signora Presidente del Consiglio, sta facendo esattamente l'opposto, nonostante il mondo intero ormai stia faticosamente comprendendo che la strada è obbligata,

L'aumento del bilancio deve servire ad aiutare le fasce di popolazione impoverite dall'inflazione. Questa esigenza, invece, è stata espunta dalla lista delle priorità anche nel dibattito sul Patto di stabilità c'è la stessa clamorosa assenza. L'equilibrio non può essere solo tra rigore e investimenti, trascurando la vita delle persone reali. Io ritengo molto grave che si parli di flessibilità solo per le spese militari e si riconosca priorità assoluta alla necessità di portare quelle spese al 2 per cento del PIL, mentre si abbandona ogni sostegno alla popolazione. *(Applausi)*. Le spese militari vanno diminuite, altro che aumentate!

Questo sarebbe il dovere di un Governo capace di mettere al primo posto non l'idea astratta di Nazione, ma la condizione materiale di chi in quella che chiamate Nazione e in tutta Europa ci vive e anzi fatica sempre di più a viverci. *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente del Consiglio, onorevoli Ministri e Sottosegretari, colleghi, io mi aspetterei ogni tanto qualche titolo positivo da qualche giornale di quelli che annunciano sempre la catastrofe del Governo, la sciagura della Meloni - fanno addirittura i libri - e la spaccatura della maggioranza. Oggi lei, Presidente del Consiglio, ha ricordato cose che non dice lei o che non dico io, che arrivo buon ultimo, ma che dicono l'Istat e la realtà della storia. Partiamo quindi dai fatti, dai titoli che si potrebbero fare sui giornali anche descrivendo questo dibattito: PNRR, ok a tutta una serie di rate. Sono cifre ingenti che sono state erogate correggendo gli errori fatti dai Governi del passato, i cui piani sono stati respinti a livello europeo. se nottetempo Di Maio mandava le note che la presidente del Consiglio Meloni prima ha citato, di giorno Conte mandava piani sul PNRR che sono stati rimandati indietro. Non ha neanche scelto le tenebre. Questo Governo ha rimesso a posto le carte, ha negoziato con fatica. C'è qui il ministro Fitto - lo conosco da troppo tempo per essere considerato un adulatore dell'ultimo minuto - che fa un lavoro politico serio, istituzionale. E, a volte, anche noi dobbiamo comprendere che, per convincere un po' di eurocrati, bisogna essere anche un po' più flessibili su questioni che pure riteniamo vedano l'Italia avere ragione. Questo è il dato. Le promozioni delle società di *rating* sono un fatto o sono una manipolazione delle forze oscure del centrodestra? Promozioni su promozioni per un Paese che ha un debito pubblico gigantesco, storico, che si è formato nel tempo e, quindi, rende più faticoso l'esame. Siamo come una classe di una scuola che subisce sempre un po' di pregiudizio da parte dei professori, per un accumulo storico non riguardante questo Governo: è un dato di fatto che, insieme all'andamento del PNRR, rivendichiamo. La riscrittura delle direttive europee sballate per colpa della sinistra la sta ottenendo il fronte moderato europeo; è il Governo italiano che l'ha chiesto, sono i nostri Ministri e anche il Partito Popolare Europeo. La casa e l'automobile non si possono cambiare domani mattina,

alternative alla sinistra possano governare l'Europa senza confusioni e senza commistioni. Quelle che fanno parte di questo Governo, Forza Italia nel PPE, Fratelli d'Italia e la Lega, sono forze tutte compatibili con una storia e una cultura di Governo. Quindi, siamo noi che stiamo facendo riscrivere le direttive europee sbagliate e il prossimo Parlamento europeo e la prossima Commissione lo faranno ancora più energia. Forza Italia fa dell'energia nucleare e delle centrali nucleari una priorità, perché più energia vuol dire meno povertà, più lavoro, più indipendenza. Non dobbiamo inseguire un giorno i russi e un giorno gli algerini, visto che i buoni di oggi potrebbero essere i cattivi di domani: la storia è mutevole.

dipenda dall'imbrattamento dei monumenti e dall'inquinamento del Canal Grande. Noi da questi ambientalisti da operetta non ci facciamo impressionare, visto che non difendono né l'ambiente né il futuro. Questa è la realtà che vogliamo qui enunciare e questo fa parte dei programmi europei. Quanto all'economia,

C'è una maggiore omogeneità fiscale e l'Europa deve avere più coraggio. È stato il Governo di centrodestra ad anticipare la *web tax* sui colossi della Rete, che l'Europa rinvia sempre, inginocchiandosi troppo davanti a Google, ad Amazon e ad altri. Questo Governo sta tentando di far pagare le tasse a chi non le paga. Questo non è stato fatto dai Governi del passato, che ai giganti della Rete forse chiedevano qualche cortesia o qualche favore. L'Europa deve essere più coraggiosa: se la ricchezza si sposta nel digitale, le aziende del digitale non possono essere esentasse, mentre l'ultimo commerciante o artigiano pagano per tutti. Abbiamo chiesto la riduzione dei tassi

Meloni, lei con Macron ogni tanto si incontra. Oltre a dire chi deve essere il prossimo Presidente italiano della Commissione europea - cosa che già è un'ammissione di incapacità della Francia, che lo poteva cercare tra i cittadini francesi e invece lo viene a cercare in Italia e a Roma - Macron faccia una telefonata alla Lagarde, che è francese, e le dica di

non abbiamo una visione fobica del MES, ma ci vuole un controllo delle istituzioni democratiche europee. Non ci può essere un'istituzione che non risponda al Parlamento europeo. Noi vogliamo, come PPE e come Forza Italia, che ci sia democrazia anche nel controllo di nuovi strumenti. Poi ne discuteremo, ma con il Patto di stabilità, con l'unione fiscale, con l'omogeneità delle normative bancarie e di altri settori. Non si discute solo un capitolo: si scrive tutto il libro dell'Europa del futuro e poi si vedrà anche questo capitolo così delicato e controverso. Credo quindi che quanto da lei detto vada ribadito.

decresce e dimostra che la politica assistenzialista del reddito di cittadinanza ha favorito non l'occupazione, ma solo una politica clientelare e assistenziale che ha mortificato chi lo prendeva e vuole un lavoro. Questo Governo crea condizioni perché si realizzi lavoro produttivo e non assistenzialismo.

che la Presidente del Consiglio ha evocato e alla quale devo dire anche il ministro degli esteri Tajani ha dedicato tanta attenzione in questo primo anno di Governo. Con i Balcani c'è una storia complicata di guerra e di conflitti che oggi marcia verso un'integrazione europea e una politica dell'allargamento dalla Bosnia-Erzegovina ad altre realtà. Pensiamo ancora alla difesa europea, un capitolo da scrivere che va incrementato, e al tema dell'immigrazione. Non tutti gli immigrati sono aperti al fondamentalismo. Nessuno l'ha mai detto. Questo Governo ha fatto flussi di ingresso per 400.000 persone più in tre anni: molto, direi. Ci sono poi controlli per sapere chi viene, dove va, se è dedito anche a un orientamento fondamentalista. Io mi sono stancato di vedere al telegiornale accoltellato Tizio e Caio e, dopo due minuti, si sa la biografia perché erano persone conosciute, radicalizzate, alle quali

due popoli, due Stati. I popoli sono due, il popolo palestinese e il popolo israeliano. Peccato che gli Stati non siano due. Lo Stato di Israele è uno Stato democratico, dove si è votato tantissime volte negli ultimi anni, e l'unica democrazia nel Medio Oriente, come si ricorda spesso in mezzo a monarchie, satrapie e quant'altro. Il popolo palestinese è un popolo. Ma, mentre lo Stato di Israele ha uno Stato, Hamas non è lo Stato del popolo palestinese. *(Applausi)*. È una congrega di terroristi e assassini. Non è uno Stato! Non è uno Stato! Quel popolo si liberi da una parvenza di Stato, di fondamentalisti e di assassini. Ma le avete viste le immagini di orrore, quelle che circolano e quelle che a volte anche le televisioni hanno ritegno di mostrare, con donne stuprate e sgozzate? Siamo tutti sensibili alla violenza sulle donne e mi pare strano che alcuni si dimenticano le donne e le ragazze israeliane sequestrate, stuprate e uccise, come se non fossero fossero donne come le ragazze italiane o di qualsiasi Paese vittime di violenze... ...Due Popoli e due Stati, ma al momento all'appello rispondono due popoli e uno Stato. Speriamo che l'altro Stato nasca e non nel segno di Hamas, del suo terrorismo e della ripresa di antisemitismo che anche lei ha denunciato. Faremo quindi la nostra parte in Europa, sapendo che molto c'è da fare, che il debito pubblico è grande, ma che senza gli sprechi dei Governi Conte, senza gli errori di una politica demagogica, l'Italia viene apprezzata in Europa, per il PNRR, dalle società di *rating* e per tutti gli altri sforzi che anche con la legge di stabilità nelle prossime ore faremo. Qualcuno si occupa dell'elemosina parlamentare: noi ci occupiamo dei contratti del pubblico impiego, del taglio al cuneo fiscale, di scelte importanti che ci renderanno più forti quando dovremo andare agli altri esami europei. Gli esami non finiscono mai, ma ci sono quelli che vengono bocciati appena si presentano e quelli, come il centrodestra, che gli esami li affrontano e li superano. Per tali ragioni voteremo con convinzione la risoluzione che abbiamo sottoscritto. *(M5S)*. Signor Presidente, mi tocca ancora una volta prendere la parola dopo il senatore Gasparri, che evidentemente ancora non si è dimesso. Presidente Meloni, lo chiedo a lei: il presidente Gasparri ha ha chiarito i suoi interessi nelle commesse di Stato in ambito di cybersicurezza e con i servizi segreti di Stati stranieri? *(Applausi)*. E già che ci siamo, anche la ministra Santanchè, dopo aver mentito in faccia agli italiani, ha almeno pagato il TFR dei suoi dipendenti? L'onorevole Del Mastro è ancora al suo posto, dopo aver spifferato informazioni segretate al coinquilino, che le ha usate politicamente per attaccare le opposizioni? E l'immarcescibile Vittorio Sgarbi ha dichiarato o meno le entrate delle sue ricche consulenze? Visto che va in Europa, presidente Meloni, si faccia spiegare dai suoi omologhi europei... Visto che va in Europa, presidente Meloni, colga l'occasione per farsi spiegare dai suoi omologhi europei come gestiscono a casa loro casi simili, come si sta con disciplina e onore nei ruoli di governo di una Nazione europea. Veniamo al tema. Seguirò l'ordine degli argomenti che ha seguito lei, presidente Meloni. dalla modifica del Patto di stabilità. Lei è venuta qui a raccontare che oggi - e cito - la posizione negoziale dell'Italia parte da una base di credibilità e da una serietà che sono riconosciute alla nostra Nazione grazie al lavoro di questo Governo, in particolare grazie al lavoro del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Qual è il grande lavoro del ministro Giorgetti? Tagli, tagli e ancora tagli. *(Applausi)*. Tagli all'istruzione, tagli alla sanità, tagli al sociale, tagli alle pensioni: "Giorgetti mani di forbice" è il nuovo film di Natale. *(Applausi)*. Due manovre economiche lacrime e sangue e lei ha il coraggio di dire che, grazie a questo, si è conquistata credibilità in Europa. È esattamente il contrario: Giorgetti in Europa non sta toccando palla; l'Italia è in tribuna a guardare un *match* giocato da altri, in particolare da Francia e Germania, e il Governo dei patrioti è ridotto a fare il tifo per i francesi. E siccome sa già che non porterà a casa niente, sta facendo una novità assoluta: *austerity* preventiva, così prepara gli italiani a quando le regole soffocanti del Patto di stabilità torneranno pienamente in vigore, sperando che non si accorgano della differenza. Lei, presidente Meloni, sta facendo perdere un treno importantissimo a questo Paese, un treno che potrebbe non passare mai più. Se lei non è in grado di afferrare questo treno, presidente Meloni, provi a chiedere a suo cognato: il ministro Lollobrigida è bravissimo a fermare i treni. Ma no, presidente Meloni. Queste sono battute, ma la situazione è seria. Lei viene in Parlamento, invece, e la butta in caciara, accusando qualunque cosa piuttosto che la palese incapacità di gestione di questo Governo. Devo ricordarle, presidente Meloni, che non poco tempo fa lei aveva annunciato trionfante che la manovra economica si sarebbe chiusa entro il 15 dicembre. Oggi è il 13 dicembre e e l'esame della manovra in Commissione praticamente non è ancora iniziato. Avete anche silenziato la vostra stessa maggioranza, introducendo la "zero letture", niente emendamenti anche per le forze di maggioranza, ma il Governo si auto-emenda nottetempo, inviando pacchetti di emendamenti - quelli sì nottetempo - presidente Meloni. Allora, se la gestione della manovra economica è lo specchio della gestione delle finanze del Paese, questo rispecchia la vostra incapacità di gestire l'economia, che infatti sta andando a picco. Lei nelle sue repliche, presidente Meloni, ha citato l'Istat sull'occupazione. Peccato che si è dimenticata di citare l'Istat sul crollo della crescita, sul crollo degli investimenti, sul crollo della produzione industriale. Presidente, si rende conto che la produzione industriale è ferma ormai da nove mesi consecutivi? Si rende conto di cosa significa questo per il nostro Paese? Per negare questo fallimento in ambito economico, presidente Meloni, lei continua come una macchietta ad accusare tutto e tutti. La verità è che non c'è mai stato un Governo fortunato come il vostro; un Governo che si è ritrovato

209 miliardi che ancora non siete in grado di gestire e, per giustificare questa vostra incapacità, continuate ancora imperterriti con la balla del buco del superbonus. Allora gliela dico io, una volta buona, agli italiani la storia vera del superbonus: avete fatto tutti a gara gara - Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega - per intestarvelo con convegni, manifestazioni, emendamenti; avete fatto qualunque cosa per cercare di strappare la paternità al superbonus targato MoVimento 5 Stelle. Vi siete fatti eleggere al grido di «difendiamo il superbonus». Quando poi vi siete resi conto che questa operazione era fallita e che la paternità del provvedimento, che era stato lodato anche dall'Europa, rimaneva in capo al MoVimento 5 Stelle e a Giuseppe Conte, avete deciso che andava demonizzato. E così avete demonizzato il superbonus per distruggere il MoVimento 5 Stelle, fregandovene delle conseguenze sulle famiglie, sui condomini e sugli imprenditori onesti. *(Applausi)*. Questo è quello che siete stati disposti a fare. fare. Vede, Presidente, voi, più di chiunque altro, sapete bene che purtroppo la propaganda fa più consenso dei fatti e ne fate un uso cinico, perché lei, presidente Meloni, sarà credibile nel parlare dei soldi degli italiani quando avrà lasciato un PIL al 7,4 per cento, come abbiamo fatto noi con il presidente Conte. Lei sarà credibile quando avrà messo a terra qualche progetto del PNRR, invece di perdere 16 miliardi destinati alle periferie, alla sanità e agli asili nido. *(Applausi)*. Lei sarà credibile quando manterrà gli annunci sugli extraprofitti delle banche. «Andremo dritti», aveva detto dritti come un'inversione a U. L'ha detto poco fa, l'ha riconosciuto lei stessa: le banche hanno fatto extraprofitti enormi anche sui *bonus* edilizi. Tanto più: tassateli allora. Invece, continuate a tartassare i poveracci e bocciate il salario minimo. Glielo dica ai suoi amici in Europa che lei ha bocciato il salario minimo in Italia, quando loro hanno tutti il salario minimo. una nobile battaglia in Europa la sta conducendo, Presidente, e si sta battendo come una leonessa: questo glielo riconosciamo. Si sta battendo per lo scorporo delle spese militari dal Patto di stabilità e su questo c'è un ampio consenso in Europa, per cui ci avete puntato una bella *fiche*, così sperate di prendere due piccioni con una fava. Vi intesterete l'eventuale successo di questo bel merito ricompenserete i veri grandi *sponsor* di questo Governo: le *lobby* delle armi. Il motto di questo Governo è «più armi e più guerra per tutti» *(Applausi)*. È un Governo bellicista e guerrafondaio. Però, Presidente, lei la deve smettere di mentire, come ha fatto anche poco fa in Aula. Se Conte ha firmato commesse di armi destinate a Israele, lo ha fatto quando Israele non era entrato in guerra con una Palestina che non esiste. Allora piuttosto ci dica, visto che dice di aver fermato le commesse, ha fermato anche quelle in essere? Non scappi e risponda ad una semplice domanda. Infine, chiudo sul MES,

Presidente del Consiglio, se non lo vuole ratificare, è libera di non farlo, è lei che decide, si assuma le sue responsabilità. Sa perché ha paura? Perché sul Patto di stabilità non avete ottenuto nulla; altro che logiche di pacchetto. Per questi motivi e per tutti quelli che non ho potuto elencare per mancanza di tempo, il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, voterà decisamente no alla risoluzione di maggioranza.

Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega alla risoluzione della maggioranza e alle risoluzioni su cui il Governo ha dato parere favorevole.

giusto che il Governo italiano abbia confermato l'impegno nei confronti dell'Ucraina in relazione a tutti i suoi aspetti e ci permettiamo di dare un piccolo suggerimento, visto che comunque le parole hanno decisamente un peso. Suggeriamo di non parlare solo di pace giusta, perché, se cominciassimo a entrare nell'ottica anche di una pace possibile, tutta Europa, a nostro giudizio, farebbe un passo in avanti, senza confondere aggressore con aggredito, senza fotografare indubbiamente la realtà attuale, che significherebbe sostanzialmente una resa. resa. Non possiamo però neanche continuare a sostenere che la pace sia possibile solo se la Russia si ritira e se comunque viene sconfitta a livello militare, perché sostenere questo significherebbe continuare la guerra all'infinito con tutte le sue conseguenze e che non vi sia invece la vera possibilità di trovare una soluzione di carattere diplomatico. In Medio Oriente, Israele giustamente deve respingere e rispondere agli attacchi del 7 ottobre, come abbiamo più volte sostenuto in quest'Aula, ma deve dare una risposta intelligente e non radicale:

ogni iniziativa possibile per la liberazione degli ostaggi ancora detenuti e naturalmente proteggere anche i civili di Gaza.

non solo alla tematica e alla discussione relativa al suo possibile ingresso nell'Unione europea. Pensate anche a diversi Paesi arabi e al Medio Oriente, le cui agende non sono più compatibili con Hamas e con i terroristi. Avete visto anche l'esempio dell'Arabia Saudita, *in primis*, e il fatto che si cominci a guardare agli scambi commerciali, alle relazioni internazionali, al turismo (dimostrazione ne è Expo 2030) e al mondo del calcio, per fare alcuni esempi che vanno nella direzione di un mondo arabo che vuole aprirsi a una realtà diversa e comincia a reputare il terrorismo un problema per lo sviluppo economico di quei territori. La forza dell'economia: è questa allora la strada che bisogna perseguire, se vogliamo ottenere risultati che vadano verso il superamento di questi conflitti, di questa estrema conflittualità, di un mondo sempre in competizione e di queste guerre che stanno generando instabilità nei mercati e difficoltà per tutta la popolazione mondiale alle varie latitudini. Sulla *governance* europea, in conclusione, è giusto ridurre il debito e il disavanzo eccessivi. Questo è un dovere che ogni Stato deve portare avanti. Però bisogna fare attenzione a vincoli troppo stringenti e a percorsi di aggiustamento troppo rigorosi, fondamentalmente impossibili da mantenere, che rischiano di causare danni irreparabili alla nostra economia e alla nostra società, anziché generare benefici. Bisogna invece puntare, come sottolineiamo noi, sulla valorizzazione degli investimenti, soprattutto sul tema della transizione energetica e digitale. Se si penalizzano gli investimenti, come qualcuno in Europa vuole fare, è difficile pensare che l'Eurozona possa crescere. Questa vecchia Europa, Questa vecchia Europa, se non comprende, rischia davvero di essere perduta. Questo è il messaggio che dobbiamo dare noi

sui mercati, in realtà è sostenibile data l'elevata capienza del risparmio privato. Paolo Savona, Presidente di Consob, di recente ha detto che il risparmio italiano è largamente capiente per accogliere l'indebitamento pubblico

dove ognuno deve recitare la sua parte anziché mettersi a ragionare e questa, forse, è la notizia più sconfortante per la politica attuale in generale di tutto l'arco costituzionale, lo dico per esperienza. Ciò detto, io sono tra i principali sostenitori della *Realpolitik*, che è fatta di ottimi rapporti internazionali, senso delle istituzioni, giusti equilibri, atlantismo, e penso che questo Governo sotto tale aspetto si stia muovendo benissimo, anzi addirittura sia arrivato a spiazzare l'opposizione.

veda nelle banche italiane una ricca preda da conquistare, essendo un giacimento di risparmio tra i più ricchi d'Europa. Per noi della Lega il risparmio degli italiani viene al primo posto, è un messaggio molto chiaro che diamo agli oligarchi di Bruxelles.

Nel 2020 è andata esattamente così: di fronte alla pandemia, al crollo dell'economia, l'Europa ha avuto il coraggio di fare il salto di qualità che era necessario, fino a Next generation EU. È stata una risposta all'altezza delle sfide che avevamo di fronte, perché c'era una classe dirigente, in Italia e in Europa, che si è assunta le proprie responsabilità e che ha saputo immaginare e costruire quel cambio di passo che era necessario. uno degli esponenti più importanti di quella classe dirigente, un italiano coraggioso che ci ha lasciato prematuramente, David Sassoli. Presidente, negli ultimi tre anni abbiamo dovuto fare i conti con più crisi sovrapposte: la crisi energetica, l'inflazione, le crisi geopolitiche, i nuovi rapporti di forza a livello internazionale, la doppia transizione. Ora, l'attuale classe dirigente, di cui Giorgia Meloni fa pienamente parte, deve decidere quale ruolo l'Europa vuole svolgere in questa fase della storia mondiale, se un ruolo da gregaria o da protagonista, e deve deciderlo innanzitutto sul piano geopolitico. Mario Draghi, quello della foto, Presidente, ha detto pochi giorni fa parole che condivido: l'Europa in una fase critica deve unirsi e deve diventare uno Stato. Questa è la prospettiva: gli Stati Uniti d'Europa. Noi stiamo da quella parte, voi state dalla parte dell'Europa minima, come ha detto anche oggi la presidente Meloni. *(Applausi)*. La guerra in Ucraina, dal punto di vista geopolitico, rimane il banco di prova più importante. Siamo in una fase delicatissima. Presidente, la posizione del Partito Democratico non è cambiata, anzi, questo è a maggior ragione il momento di tenere il punto, di garantire tutte le forme di assistenza necessarie per assicurare il diritto di autodifesa dell'Ucraina,

una pace ingiusta e fondata sul sopruso non è pacificazione, ma usurpazione che promette di far finire la guerra, ma segna l'inizio di un'epoca di instabilità, con i *leader* autoritari autorizzati fin dal primo giorno a sostituire il diritto con la forza. Noi non vogliamo vivere in quel mondo, ma allora dobbiamo essere coerenti e conseguenti, perché questo, signor Presidente, non è il tempo dei due piedi in due scarpe; è il tempo di scegliere se stare dalla parte del popolo ucraino, oppure da quella dei sovranisti, dalla parte di Zelensky o di Orban, dalla parte del presidente Biden o dei repubblicani americani che stanno bloccando gli aiuti all'Ucraina. *(Applausi)*. Dobbiamo scegliere se essere a favore della proposta di riforma dei trattati votata dal Parlamento, che va verso un'Europa più incisiva, oppure se stare dalla parte dell'Europa minima, che fa poco o niente, come vogliono i sovranisti. *(Applausi)*. Nel Consiglio europeo, signora Presidente del Consiglio, si discuterà anche della seconda crisi geopolitica che è esplosa con la barbara aggressione di Hamas del 7 ottobre. Noi esprimiamo anche in questa sede la più netta condanna dell'aggressione dei terroristi di Hamas, la vicinanza verso il popolo israeliano, la condanna dei rigurgiti di antisemitismo e la riaffermazione del diritto di Israele ad esistere come Stato in pace e in sicurezza. il diritto sacrosanto di autodifesa non può e non deve travalicare mai il diritto internazionale ed umanitario e io credo che le parole del presidente Biden, che ha detto che Israele sta cominciando a perdere il sostegno in tutto il mondo, debbano fare riflettere fare riflettere Israele, la sua classe dirigente e gli amici di Israele in tutto il mondo. È per questo motivo che noi nella nostra proposta di risoluzione invitiamo il Governo italiano a sostenere la richiesta di un cessate il fuoco umanitario. Dobbiamo fermare i bombardamenti, dobbiamo lavorare per liberare gli ostaggi, dobbiamo garantire gli aiuti umanitari per i civili palestinesi e lavorare per il dispiegamento di una forza di interposizione. Dobbiamo lavorare, soprattutto, per per riaprire una prospettiva di pace e di coesistenza, perché due popoli e due Stati non deve rimanere uno slogan, ma deve essere un obiettivo politico verso cui l'Europa deve tendere. del Consiglio, si confronterà anche sulla riforma della *governance* economica. Il vecchio Patto di stabilità ha mostrato tutti i suoi limiti: non ha garantito né la stabilità dei conti, né tantomeno la crescita economica e fa sorridere il concetto che emerge nel dibattito secondo cui sarebbe meglio ritornare alle regole che in dieci anni hanno significato l'austerità per il nostro Paese. La Commissione europea aveva presentato una proposta che affrontava molte delle criticità delle vecchie regole: la prospettiva pluriennale anziché di breve periodo, variabili osservabili anziché quelle che erano al centro del vecchio Patto; piani costruiti sulla base delle specificità dei singoli Paesi. Non era il migliore dei mondi possibili, signora presidente del Consiglio Meloni, ma rappresentava un passo in avanti. Il problema è che i negoziati tra i Governi nazionali ci stanno portando in una direzione molto diversa dalla proposta della Commissione, perché nelle bozze che stanno circolando tornano le regole di riduzione del debito e soprattutto le regole automatiche di riduzione del *deficit* e sono regole stringenti per un Paese come l'Italia. Sono regole automatiche e procicliche, che valgono anche quando l'economia va male.

non sarà certo la gentile concessione di tre anni di ammorbidimento di regole a cambiare il quadro, perché il quadro è il ritorno dell'austerità in Europa e c'è di cosa essere molto preoccupati per come stanno andando le cose. Voi vi eravate illusi e avevate illuso il Parlamento che la mancata ratifica del Trattato MES potesse essere utilizzata come merce di scambio per avere un quadro più favorevole all'Italia. Ce lo dobbiamo dire, Presidente: la pantomima sul MES ha indebolito, non ha rafforzato la posizione dell'Italia. Per anni avete raccontato che il MES era un cappio per l'Italia - questa era la propaganda di Fratelli d'Italia e della Lega - ma nel frattempo il Trattato veniva ratificato quindi da Governi di sinistra e Governi di destra, Paesi ricchi e Paesi meno avanzati, grandi Paesi e piccoli Paesi. Manca solo l'Italia. Manca solo l'Italia. Capisco che sia difficile di fronte ai propri elettori rimangiarsi anni di *slogan*, di *post* sui *social*, di propaganda, di promesse elettorali. Però lo avete già fatto: vi siete rimangiati le promesse sulle pensioni e le promesse sui migranti, e lo dovrete fare anche sul MES. Se ne faccia una ragione, presidente Meloni,

il 9 dicembre del 2020 il Parlamento della Repubblica italiana ha invitato il Governo a finalizzare l'accordo sul Trattato MES e il voto in quest'Aula è avvenuto con 156 voti a favore, 129 contrari e quattro astenuti. Questa è la storia. Altro che favore delle tenebre: c'è stato un voto del Parlamento italiano. Lasci perdere la propaganda e le tenebre, signor Presidente del Consiglio, e confrontiamoci a viso aperto. L'austerità cieca che era uscita dalla porta, perché noi avevamo fatto Next Generation EU, rischia di rientrare dalla finestra, anche perché non avete fatto valere fino in fondo il peso dell'Italia. Del resto, è stato già detto e diciamocelo: l'austerità è già tornata in Italia, perché la legge di bilancio, che noi cerchiamo di discutere *(Applausi)*, taglia le pensioni, non mette un euro sulla casa, non mette un euro sul trasporto pubblico e riduce la spesa sanitaria in rapporto al PIL, che è l'unico indicatore serio da prendere a riferimento. Siamo di fronte a un bivio, signor Presidente, e con l'ideologia sovranista, andando a braccetto con Orban e con Abascal, l'Italia finisce su un binario morto, in un vicolo cieco. La presidente Meloni ha detto che vogliono essere pragmatici. Noi sul pragmatismo ci siamo, ma fatelo veramente e non a chiacchiere, perché sta a voi portare il Paese nella direzione giusta.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, innanzitutto voglio sottolineare che la presenza del Presidente del Consiglio e

ed era la terza volta che accadeva negli ultimi dieci anni: questo è un fatto significativo. Anche i Ministri hanno dimostrato la loro presenza. Questo quando si parla del ruolo

cosa che non si può dire di colui che ci ha accusato di fare da mera *claque*. Non ne faccio il nome, ma dico che è stato sindaco di Firenze e nel passato anche Presidente del Consiglio;

maggior parte del tempo non c'è stato visto che era in corso un'importante partita di calcio, che peraltro andò pure male per la nostra Nazionale. Il Consiglio europeo vedrà l'Italia con un ruolo centrale e da protagonista, nonostante qualcuno forse speri che ciò non avvenga. Questo per una serie di ragioni: per la capacità del presidente Meloni, con l'intero Governo, come lei ci ha riferito e cosa per la quale viene anche criticata, di saper parlare con tutti. L'Europa ha 27 Paesi membri; ne sono di molto grandi e molto importanti, come la Germania, la Francia e l'Italia, altri più piccoli, altri piccolissimi, ma poi votano tutti quanti e bisogna avere rapporti con tutti perché non scegliamo noi, ma i cittadini degli altri

degli interessi comuni con i grandi Paesi europei, su altri invece possiamo avere argomenti in comune con altri ancora. Questo è uno degli aspetti. Un altro aspetto è il fatto di avere un Presidente del Consiglio che sarà tale per i prossimi anni perché ha avuto un chiaro mandato dagli elettori, perché c'è una coalizione unita e coesa e perché è espressione diretta del voto dei cittadini. Parliamo per esempio dei sindaci, del governo delle nostre città; ci sono stati dei commissari, evidentemente non votati, persone stimabilissime, di prestigio, vice prefetti e così via, ma chi fa la politica e chi viene davvero ritenuto un rappresentante di una città è colui che viene eletto, indipendentemente dal prestigio di chi sia il commissario che non discutiamo. A livello internazionale il fatto che il nostro Capo del Governo sia espressione dei cittadini è un aspetto molto importante e la riforma del premierato fa

capacità di relazionarci con tutti ci ha consentito a livello europeo di ottenere degli importanti risultati, ad esempio, sull'euro 5, dove il rischio era che centinaia di migliaia, milioni forse di automobilisti italiani, non potendosi permettere l'auto nuova, non potessero più circolare subito o nel breve periodo. Pensiamo ancora alle case *green*; ci sono state delle dilazioni ragionevoli per fare in modo che questa transizione, alla quale qualche collega dell'opposizione ci ha richiamato, sia ecologica e non e non ideologica, dove indipendentemente dal risultato sull'ambiente bisogna imporre determinati modelli ai quali magari non si è pronti. *(Applausi)*. Parlo, per esempio, dell'elettrico, della rete, del del fatto che in Italia non c'è neanche un impianto. Quando è iniziato il lavoro di questo Governo, non c'era neanche un impianto per lo smaltimento del litio, cosa fondamentale perché poi anche le batterie si esauriscono esauriscono e dunque occorre intervenire. Vi è poi un altro aspetto che dà prestigio e forza alla presenza italiana a livello europeo e internazionale: il fatto di aver avuto dei risultati economici

nel corso del 2023 ha avuto la media di 176 che, tra l'altro, guarda caso, è proprio il livello che c'è oggi, rispetto a 196 che è stato il livello medio del 2022. Non è quindi un fatto episodico, legato magari ai picchi che si videro nel mese di settembre dell'anno scorso,

non per avere magari qualche aspetto che possa interessare per fare qualche spesuccia elettorale in più, ma per avere un'Europa che punta allo sviluppo e alla crescita e non ad una ad una cieca austerità. È curioso che ci venga rimproverata dall'esponente del MoVimento 5 Stelle questa presunta austerità: è un'austerità dove l'occupazione raggiunge livelli *record* storici. Ad averne di austerità! Il fatto è che non è austerità: è aver saputo concentrare le risorse su ciò che serve all'Italia e su ciò che serve agli italiani, per stimolare l'occupazione e la crescita, anziché perdersi tra mille rivoli di bonus, superbonus

comprati a centinaia di migliaia a prezzi superiori rispetto a quelli che si potevano trovare tranquillamente su Internet, comprandone uno solo. *(Applausi)*. Questo è un mistero nelle capacità negoziali di condurre determinati tipi di acquisti. quando si parla di austerità, se c'è la necessità (e c'è stata) di limitare gli interventi, avremmo voluto ridurre ancora di più le imposte ai redditi medio-bassi, avremmo voluto aiutare ancora di più le famiglie sulla natalità (più ancora di quanto viene

che tutte le truffe siano state scoperte (evidentemente ce ne sono delle altre), è evidente che si è dovuto fare una finanziaria prudente, concentrando le risorse. 20 miliardi equivalgono a circa 850 euro per ogni italiano che lavora, in un anno. È chiaro che, se ci fosse stata questa somma a disposizione, avremmo potuto agire in modo ben diverso. Sorprende anche sentir parlare di spese per le armi,

europea nel difendere gli interessi di tutti gli italiani, che lei rappresenta.

nn. 9, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 26, mentre ha espresso parere favorevole con riformulazioni accettate dai presentatori sugli impegni nn. 3, 5, 11 e 14. Il parere è favorevole sui restanti impegni. Il senatore Alfieri ha chiesto la votazione per parti separate. Metto ai voti la proposta

migliaia di famiglie italiane. Stiamo parlando dei disabili, degli *over* 60 e di famiglie con bambini che dal prossimo anno vedranno il passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione,

per ricevere questo sussidio già dal mese di gennaio, come previsto dalla legge. *(Brusio).* Purtroppo, il Governo è in forte ritardo,

purtroppo sta facendo un regalo di Natale a tutte le famiglie con disabili o *over* 60, quelli che sono stati definiti non occupabili dal meccanismo che supera il reddito di cittadinanza, ossia l'assegno di inclusione. Secondo quanto previsto da questo Governo, avrebbe già dovuto esserci una piattaforma dedicata sul sito dell'INPS dove i beneficiari, già in questo mese, che è l'ultimo in cui percepiscono il vecchio sussidio del reddito di cittadinanza, avrebbero dovuto fare domanda per ricevere il nuovo contributo, l'assegno di inclusione, già dal prossimo anno. Tutto questo, purtroppo, non è accaduto, infatti i decreti attuativi sono in forte ritardo e se non vengono emanati non avremo nemmeno la piattaforma sulla quale i beneficiari potranno fare la domanda. comporterà per queste famiglie che sono in un gravissimo stato di disagio sociale un bel regalo di Natale. Questo Governo, quindi, continua a fare cassa sui più fragili, sui più deboli, continua ad essere

quindi arrecando loro un danno gravissimo, perché stiamo parlando di famiglie che non hanno da vivere o che hanno delle gravissime disabilità, dei gravissimi drammi di salute al proprio interno

anche quando non sono l'unica a parlare in quest'Aula, lei mi riprende con una certa severità. Passi quando me lo merito, ma se parliamo in dieci e lei punta il dito contro di me esclusivamente, mi sembra una questione personale. Capisco che ho un tono di voce particolare, ma oggi ho appositamente abbassato la voce proprio per evitare le sue rimostranze, che però puntualmente sono arrivate. Capisco che alla maggioranza dia fastidio che qualcuno si indigni quando vengono fatte determinate osservazioni, ma anche quando sono pacate mi pare veramente assurdo, soprattutto perché è normale che l'opposizione si indigni quando in quest'Aula si cerca di spacciare per verità assolute delle clamorose bugie, come è avvenuto quest'oggi con la presidente Meloni che parlava del finanziamento sul Fondo sanitario nazionale. Per le bugie io mi indigno sempre, cercherò di farlo con meno veemenza, ma chiedo a lei se per caso la sua puntualità nel riprendere me non sia dovuta, più che al mio tono di voce, al fatto che io sia una donna e quindi spicco di più tra gli altri.

però, se vuole essere cortese, riguardi i video, non solo quello di oggi ma in genere di molte sedute. Se vuole le faccio fare una raccolta. Capirà, in Sicilia... *(Commenti).* No, adesso non c'è un dibattito.